Comunico che in data 18 aprile 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

rapidamente in Parlamento a riferire su quanto accaduto ieri all'istituto per minori Beccaria.

suscitato raccapriccio. Non trovo altre parole. Parliamo di un istituto per minori, che dovrebbe essere ancora di più votato alla rieducazione, nel quale sono accaduti veramente fatti dell'orrore: violenze, tentata violenza sessuale, tortura e poi lesioni aggravate. Ci sono stati arresti di 12 o 13 agenti di Polizia penitenziaria e altri otto sono stati sospesi. Già da tempo il tempo il senatore Mirabelli e la senatrice Malpezzi avevano acceso fari su questo istituto dove erano accaduti altri fatti. Il Ministro deve venire a riferire quanto prima. Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo una cosa. Ieri - è stata una casualità - i parlamentari del Partito Democratico hanno visitato circa 40 carceri in tutta Italia. Il film visto è il solito: condizioni ai limiti dell'umano in molti casi, mancanza di spazi, sovraffollamento, mancanza di agenti di Polizia penitenziaria, restrizioni nelle aperture delle sezioni con situazioni di grande tensione, non più vigilanza dinamica, mancanza della videosorveglianza. un caso: ieri i due senatori che sono dietro di me, la senatrice D'Elia e il senatore Sensi, sono andati a Regina Coeli; poco dopo hanno appreso che lì c'era stato l'ennesimo quotidiano suicidio di un detenuto. Mentre io ero a

difficilissimo, spesso in condizioni di scarsa retribuzione, ma soprattutto in condizioni difficilissime, perché sono pochi rispetto alla popolazione che sta dentro le carceri. dell'istituto Beccaria venga immediatamente a riferire il Ministro, ma in generale il Governo si sbrighi: la situazione delle carceri è davvero esplosiva e un Paese civile non può simile stato di cose, perché applicare l'articolo 27 della Costituzione significa concepire la pena come rieducazione. E, quando un detenuto che sconta una pena in carcere esce rieducato, riabilitato, formato e trova un lavoro,

Signor Presidente, le notizie che ci giungono da Milano, relative a delle denunciate, presunte violenze che sarebbero state compiute ai danni di ragazzi minorenni detenuti all'interno del carcere Beccaria da parte di agenti della Polizia penitenziaria impongono, a giudizio del Gruppo Italia Viva - il Centro- RenewEurope, una immediata iniziativa in sede parlamentare da parte del Governo e del ministro Nordio. Di per sé è sicuramente inaccettabile l'idea che soggetti che appartengono alle istituzioni statali possano avere torturato delle persone che dovevano essere trattenute in loro custodia. E rispetto ad esse non possono mai, in alcun modo, venir meno i diritti e le garanzie assicurati dal nostro ordinamento rispetto al modo con il quale anche e soprattutto i detenuti devono essere tenuti, ossia in una condizione dignitosa, umana, in una condizione di assoluto rispetto delle prerogative sancite non solo dalla legge, ma anche dalle logiche umane. Non vi è dubbio, quindi, che occorra innanzi tutto aprire una discussione in sede parlamentare, parallelamente rispetto alla competenza della magistratura, che deve seguire il proprio corso e non deve essere sovrapposta. Questa è anche la spia di una situazione che all'interno delle nostre carceri si sta sviluppando e porta a dei punti di caduta che rischiano di ingenerarsi in situazioni di drammaticità.

utilizzare la vicenda per approfondire tutte le tematiche che, nel corso delle ultime settimane, nostri colleghi parlamentari hanno sollevato con delle visite presso le strutture carcerarie e nei cui confronti continuano a vedere inevase sollecitazioni, proposte e richieste. È questa, quindi, signor Presidente, alla luce della situazione alquanto preoccupante, che getta un'ombra inquietante che deve essere assolutamente fugata, la nostra richiesta.

Nella seduta di questa mattina, dopo una serie interventi nel corso di una discussione anche approfondita sul tema, la Commissione ha preso atto, anche alla luce del numero degli emendamenti e dei tempi di calendarizzazione molto compressi, dell'impossibilità di concludere

apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, il disegno di legge n. 1110, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione,

*(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, sono certa che oggi voi, come me, stiate vivendo un sentimento di profonda ed irrefrenabile gioia. Essere oggi in quest'Aula vuol dire poter dire domani alle nuove generazioni che noi c'eravamo ed eravamo parte integrante del processo più innovativo della storia della Repubblica. Voglio complimentarmi con il Governo per averci resi per l'ennesima volta fieri di essere italiani. Stiamo mostrando al mondo il significato stesso di modernità. Finalmente abbiamo risolto il problema della natalità in Italia. Da domani, finalmente invertiremo il *trend* delle nascite che nei prossimi anni ci avrebbe messo in serie difficoltà. So anche che all'INPS, dopo aver cercato di spaccare il capello per consentire a sempre meno lavoratori di pagare la pensione a sempre più pensionati, oggi tutta la dirigenza ha avuto quasi un sussulto di orgoglio misto a commozione. Sapere che riusciremo finalmente a superare i nostri cugini francesi in termini di popolazione, dopo anni in cui abbiamo perso peso a livello internazionale, è un vero e proprio sollievo. Vedo la faccia di qualche collega un po' dubbiosa, ma sono certa che siano i soliti diffidenti, i gufi, i criticoni, quelli che non vogliono bene al nostro Paese e che non comprendono appieno il concetto di Dio, Patria e famiglia. Del resto, come si fa a non comprendere che, quando la soluzione non è rintracciabile nell'intelletto, l'unica possibilità è affidarsi alla religiosità, un'intuizione trascendentale che solo Giorgia - donna, madre e cristiana - poteva avere? E allora in che modo abbiamo risolto il problema demografico? In tanti di voi se lo chiederanno, perché forse non hanno notato che, all'interno del provvedimento che si occupa della distribuzione delle risorse che il presidente Conte ha reperito in Europa, è nascosta una norma che, pur essendo totalmente decontestualizzata, rappresenta un vero e proprio punto di svolta. Credo lo abbiano fatto per rimanere umili. Ebbene, lo abbiamo fatto attraverso la costruzione di una solida riforma organica? No, di più: lo abbiamo fatto attraverso una serie di investimenti mirati a consentire alle giovani coppie di avere nuovamente fiducia nel futuro? Nemmeno, molto di più! Lo abbiamo fatto consentendo alle donne, che devono decidere se si sentono pronte nel portare avanti una gravidanza, di fruire del sostegno di professionisti affermati come psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali? No. Abbiamo già visto come è andata a finire col bonus psicologo: poco più dell'1 per cento dei richiedenti ne ha potuto usufruire. All'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Missione 6 è dedicata alla salute e contiene interventi chiari per migliorare l'assistenza sanitaria territoriale, promuovere l'innovazione e la digitalizzazione nel settore sanitario. sanitario. Mi immagino la riunione in cui, mentre si pensava le soluzioni più adeguate e coerenti all'obiettivo 6, a un certo punto un genio si alzava di scatto e, con lo sguardo fiero e gli occhi colmi di gioia, gridava: affidiamoci alla Divina Provvidenza. Sì, perché l'idea che questa maggioranza mette sul tavolo oggi è un emendamento che, oltre a farci vergognare di essere italiani moderni che vivono in un Paese laico, mortifica per l'ennesima volta le nuove generazioni e restringe i loro diritti in un religioso abbraccio. I diritti acquisiti con grande sforzo, da generazioni coraggiose, sono stati cancellati con un emendamento che ci trascina nel passato. l'ennesima riprova, ove mai ve ne fosse bisogno, di quanto sia illusoria e anacronistica la vostra azione politica. politica. Fino a quando l'operazione nostalgia si limitava a disegnare una fiamma su un simbolo, potevate risultare semplicemente grotteschi. Oggi, però, state giocando con l'identità delle persone, la fiducia nelle istituzioni democratiche e la libertà di azione dei singoli. Siete inadeguati e state disegnando, giorno dopo giorno, un'Italia retrograda, eticamente inadeguata e senza una visione. Di questo gli italiani vi chiederanno conto. Per ora, però, lo facciamo noi, chiedendovi di non oltrepassare il limite dell'umana decenza e di prendere atto dello schiaffo che state dando alle donne di questo Paese. Abbiate la decenza di fare la cosa giusta al contrario. Vergognatevi: siete il peggiore esempio possibile per i nostri giovani. Questa operazione di brutale moralizzazione all'interno dei consultori non è a favore della vita: rappresenta solo la morte del vostro intelletto.

in realtà mi ero apprestata a intervenire in questo dibattito sul PNRR su altre questioni, e cioè sulle vicende che regolano questo importante provvedimento, su cui si basano, tra l'altro, le prospettive di crescita del prodotto interno lordo nel nostro Paese

Purtroppo, però, gli accadimenti che sono avvenuti ci spingono invece ad un'altra riflessione. La prima, Presidente, la faccio cercando tramite lei di arrivare al Presidente del Senato. Noi ormai abbiamo assunto una pratica che che è oggettivamente anticostituzionale, almeno rispetto al funzionamento bicamerale del nostro Parlamento, per cui i provvedimenti sono diventati monocamerali, e cioè vengono discussi in un'unica Aula. Accade per la legge di bilancio e per il Piano nazionale di resilienza: stiamo parlando di documenti economici fondamentali per la vita del Paese, che rappresentano anche i momenti principali del dibattito parlamentare. Quando il nostro dibattito viene così compresso, vuol dire che le cose non funzionano più. Non ci ritroviamo nelle dinamiche dell'emergenza del Covid. Quella che era stata purtroppo una prassi che poteva essere giustificata durante il Covid, non lo è più oggi, perché non siamo più in una situazione di emergenza-urgenza.

prettamente di valenza economica e blindati come questo che è stato blindato alla Camera, su cui non possiamo fare niente - diventa ancora più incomprensibile la decisione della maggioranza di presentare un emendamento di modifica alla legge n. 194. Diciamoci chiaramente che, che, se non era una modifica, non si capiva perché dovesse essere presentata. Non accetti emendamenti che non hanno senso, sono pleonastici, un orpello rispetto alla nostra tecnica legislativa. Quindi, non solo è stato presentato un emendamento di modifica, ma è stato fatto in un testo blindato, in cui la Commissione di competenza della Camera, cioè la Commissione affari sociali, non ha potuto discutere neanche una virgola. Ora, io mi attengo alla forma più che al merito - ho solo otto minuti - perché la forma in una democrazia è sostanza.

cambiare e a incidere una delle norme più importanti e più delicate della nostra storia repubblicana, che nacque nel 1978 - lo ricordo - sotto il ministro Tina Anselmi, con presidente del Consiglio Giulio Andreotti e presidente della Repubblica Leone, con un movimento nella società fortissimo. Si arrivò a una mediazione, poi approvata da un *referendum* con il 68 per cento dei voti, su una questione delicatissima. delicatissima. Questa norma è talmente delicata che, ogni volta che si cerca di toccarla, ci sono delle giuste preoccupazioni, da un lato e dall'altro. Allora io mi sarei aspettata, Presidente, da un Governo che ha come *Premier* una donna e che ha tra i suoi Ministri personalità che si occupano di queste materie, di affrontarla a viso aperto, presentando una proposta di legge in Parlamento e permettendo a questo Parlamento, come nel 1978, di parlare di interruzione volontaria di gravidanza; di affrontare nel merito i cambiamenti e le trasformazioni epidemiologiche avvenute nel nostro Paese; di parlare delle donne straniere, dell'autodeterminazione e della libertà delle donne; di cosa significa oggi essere in questo Paese una madre sola e in povertà, chi ti aiuta e chi non ti aiuta; se c'è un intervento dello Stato o meno; e tante altre questioni, come il dibattito che si è aperto adesso in Europa sul diritto all'aborto. Questo è il ruolo di questo Parlamento e non ce lo possiamo fare scippare così, non ce lo possiamo fare scippare noi donne. *(Applausi)*. Ci troviamo a subire un emendamento voluto da un pezzo di questa maggioranza, senza senza dibattito, senza discussione, senza permetterci di entrare nel merito. Se io dovessi attenermi a quelle che sono le opinioni, qui parliamo di opinioni, perché la volontà, cosa fanno le associazioni, con quali protocolli entrano (se ci entrano), come sono scelte e come operano all'interno dei consultori lo sappiamo solo dalle interviste rilasciate sui giornali da esponenti della maggioranza. Non è così che si fanno le leggi. Quando una cosa esce da qui e interviene sulla carne viva delle persone, sul loro vissuto, su momenti delicati, bisogna sapere cosa accade. E noi non sappiamo cosa accade, perché l'emendamento, cambiato tra l'altro durante il suo percorso, è vago. vago. Non abbiamo un riferimento, non c'è un'indicazione: tutto può succedere. Se permettete, il modo in cui avete agito lascia adito a parecchi dubbi sulla volontà effettiva che porta avanti questo emendamento. È una questione per la quale non bisogna essere di un colore o di un altro semplicemente di sapere cosa accade nel Paese e cosa accade a una donna quando entra in un consultorio in Italia, con l'intenzione di accedere all'aborto.

intervenivate con i servizi alla persona, con una nuova legge, che in Italia non c'è, per le ragazze madri; con un sostegno, come avviene in Francia. Intervenivate con queste misure e non con un'azione che, sinceramente, ha ha tutto l'aspetto di una norma feticcio, di una bandiera ideologica. Ma l'ideologia di chi, di che cosa? Ma veramente pensate che una donna entra in un consultorio felice, quando si appresta a vivere uno dei momenti più drammatici della propria vita? O forse ha bisogno che nel consultorio ci siano dei professionisti, delle professionalità interdisciplinari, pagate dallo Stato, delle persone che rappresentano le istituzioni, che le diano una mano e la aiutino nel momento della sua scelta, senza giudicarla, senza farle pressioni, senza intimidirla? Queste sono le garanzie che tutte le donne vogliono. Finisco il mio intervento chiedendomi se le donne di centrodestra, che hanno votato l'attuale maggioranza e questo Governo, si aspettavano ciò. Veramente pensate che il mondo sia così? Pensate che le ragazze di vent'anni, trent'anni o quarant'anni siano così? Credete che pensano che fate bene a togliere la gratuità della pillola anticoncezionale? Invece di parlare alle ragazze dei problemi che ci sono, di aiutarle nella prevenzione rispetto alla consapevolezza di una scelta e a tutelare La prego di concludere, senatrice possibilità. Sono convinta che negli scranni della maggioranza tante persone più moderate e più equilibrate avrebbero voluto trovare una soluzione in cui noi donne eravamo tutte unite, e non separate come siamo oggi in questo Parlamento e come ci avete separato voi.

possono passare sottotraccia, ma meritano evidentemente una sottolineatura per la loro funzione, che secondo me è assolutamente strategica. Mi riferisco, ad esempio, alle disposizioni relative al potenziamento dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, un'istituzione cardine per la difesa difesa dalle minacce ibride, in particolare in questo momento di incertezza internazionale e con uno scenario politico assolutamente complicato e in continuo mutamento.

Si evidenzia che le attività cibernetiche ostili, condotte contro assetti informatici che noi riteniamo siano rilevanti per la sicurezza nazionale, hanno riguardato in particolare infrastrutture informatiche riferibili a soggetti privati, concentrando le proprie attenzioni soprattutto verso quelli che vengono definiti i servizi IT, i servizi dei trasporti, quelli bancari, e verso settori assolutamente fondamentali e importanti come quelli farmaceutico-sanitari e delle forniture energetiche. Gli attacchi informatici mirati contro gli obiettivi pubblici hanno messo nel mirino in particolare le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e - anche in questo caso - alcune strutture di carattere sanitario. sanitario. Si riscopre dunque fondamentale il contrasto a queste minacce che possono essere condotte evidentemente da *hacker*. Ma non possiamo neppure sottovalutare cyberattacchi di spionaggio che siano condotti in particolare da attori statuali ostili o da gruppi cosiddetti di *State-sponsored*, condotti attraverso quelle che vengono definite azioni strutturate con l'impegno di tecniche e di strumenti particolarmente sofisticati. Ritengo pertanto che ogni decisione e finanziamento a strutture volte al contrasto di queste minacce siano una chiave fondamentale per la nostra sicurezza nazionale. Segnalo anche un potenziamento del personale dell'Agenzia industrie e difesa, settore altrettanto strategico, specie - lo ribadiamo ancora - in questo contesto e momento storico. Potrei anche parlare del finanziamento a *start up* per lo sviluppo del mercato del *venture capital*, ma anche a opere infrastrutturali anch'esse strategiche a livello comunitario e che collegano in questo caso il nostro Paese con il resto d'Europa, come i progetti che sono stati fatti per l'Alta velocità nel Nord del nostro Paese; tutti progetti di una certa importanza. Vista la loro portata storica per il nostro Paese e l'Italia, mi sento di concordare totalmente con quelle che sono state le parole, ma anche le riflessioni,

È necessario, evidentemente, ridurre la burocrazia e i relativi costi amministrativi. Anche questo è un aspetto che ritengo estremamente importante, se si vuole una effettiva messa a terra del PNRR in maniera snella e - come dicono quelli bravi - anche in forma *smart*. riflessione riguarda le tempistiche. Personalmente, io non vedrei nulla di male ad aprire un ragionamento su un'estensione dei termini e delle scadenze, considerando anche la strategicità di tali progetti. Proprio in questo senso il ministro Giorgetti ha parlato del tema all'ultimo Ecofin, ricordando come,

che vanno nella direzione di una difesa di quelli che sono gli interessi nazionali in Europa, cosa che tanti Ministri dell'economia avrebbero dovuto fare in tempi antecedenti, ma evidentemente si sono sempre profilati dietro seconde file in riunioni europee. Per cui, in conclusione, bene sta facendo il nostro Governo sul progresso del PNRR e molto positiva è la posizione che abbiamo ascoltato, anche ieri sera in Commissione, del ministro Giorgetti. È un grande auspicio che anche quest'Aula possa davvero, tutta assieme, dare il suo supporto al Ministro e a tutto il Governo in quelle che saranno le trattative, non sicuramente facili, con i *partner* europei per addivenire ad alcune contrattazioni. In questo senso ne sarebbe sicuramente rafforzata la maggioranza, ma ritengo che il posizionamento dell'Italia debba - e non possiamo dimenticarlo - essere la nostra priorità. Per cui, sarebbe assolutamente auspicabile un'ampia condivisione di questo progetto. *(Applausi)*.

La gestione del PNRR è una delle priorità del Paese; la sua attuazione è un percorso articolato, che va dalla *governance* del Piano alla realizzazione delle opere. Il provvedimento in esame è un passo in avanti importante e decisivo per proseguire con la messa a terra dei progetti, in continuità con il lavoro che il Governo sta facendo in raccordo con la Commissione europea; lavoro che ha consentito di raggiungere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che la stessa Europa ha riconosciuto. Tutto nero su bianco, inequivocabile, con una risposta a quanti continuano ad essere gufi del PNRR. È in modo particolare a loro che bisogna parlare. Oggi esamineremo e voteremo un provvedimento che non ha tagliato risorse, ma che ha effettuato una rimodulazione, proprio per perseguire, con una scelta attenta e misurata, anche quegli obiettivi i cui tempi non consentivano la conclusione entro il 2026. Ed è per questo che oggi discutiamo un decreto-legge le cui disposizioni permetteranno al nostro Paese non solo di non perdere le risorse, ma addirittura di portarne in aggiunta. L'articolo 1 del testo è il vettore normativo tramite il quale si dà attuazione alla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, proposta dal Governo Meloni ed approvata nel corso del Consiglio Ecofin dello scorso 8 dicembre. È noto il *modus operandi* adottato dal Governo, ovvero il mestiere del fare. *(Applausi)*. Ed è proprio alla luce di un'approfondita e meditata ricognizione del PNRR che sono mutati i tempi di realizzazione di alcuni punti in particolare, rendendo incompatibile con il Piano stesso una serie di investimenti e di obiettivi. Ecco perché si è scelto di sostituirli con altrettanti, che danno invece garanzia certa di attuazione. È ormai noto ed evidente che i progetti che non avevano più i parametri per essere realizzati all'interno del PNRR non sono evaporati in un nulla di fatto, ma verranno attuati attraverso altri fonti di finanziamento, costituite da risorse già presenti nel bilancio dello Stato o su fondi come quelli per la coesione territoriale, che consentono tempi di realizzazione più ampi. Ed è sempre all'interno dell'articolo 1 che il Governo ha deciso di scandire e individuare per legge, in maniera assolutamente dettagliata, le nuove coperture per i progetti che escono formalmente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e rientrano in altri fondi.

misure. Non c'è più spazio per le fantasiose ricostruzioni delle opposizioni. Gli impegni sono sacri per questo Governo ed è per questo che qualsiasi cosa sia uscita dal PNRR per legge è stata riprogrammata e sarà comunque attuata. I fatti sono inopinabili e i numeri lo sono ancor di più. È inutile raccontare falsità ad elettori di una sinistra decisamente smarrita, a tal punto da non riuscire a fare le addizioni. Basta un dato su tutti: il saldo è positivo, i finanziamenti sono stati incrementati. Molte le cose fatte, molti gli impegni mantenuti, molte le cose che il Paese aspettava e che si concretizzano con l'approvazione di questo decreto-legge. Ed è così che si disinnescano tante polemiche. Le cose fatte, dicevo, sono tante: il trattamento economico dei lavoratori impiegati negli appalti e nei subappalti non può essere inferiore a quello previsto dal contratto nazionale; si introduce negli appalti, sia in quelli pubblici che in quelli privati, l'obbligo del controllo della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Viene disposta la cosiddetta patente a punti obbligatoria per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili. È previsto lo scorrimento delle graduatorie per gli insegnanti di sostegno. Si lavora seriamente al rilancio e alla verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità con le specifiche tecniche europee e internazionali. Si lancia l'utilizzo dell'idrogeno con l'individuazione del soggetto attuatore per quanto concerne l'ex Ilva di Taranto; si procede con la proroga delle graduatorie del personale delle scuole dell'infanzia gestite dai Comuni. Queste alcune delle misure adottate a beneficio del Paese da questo decreto-legge. Purtroppo ci stiamo abituando a colpire subito e con i fatti molte delle *fake news* che queste sinistre vogliono raccontare, ma un approfondito esame del PNRR, che a breve quest'Aula approverà definitivamente, smantella qualsiasi insensato attacco ed evidenzia una gestione oculata, attenta e partecipata del Governo Meloni e della seria e competente gestione del ministro Fitto. Il PNRR è stato fin da principio un argomento per molti ostico, ma le opposizioni, a proprio uso e consumo, se lo intestano e lo demonizzano in base a cosa gli torna comodo. Chiarito che non ci sono tagli, ma riattribuzioni di risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, da italiani dobbiamo essere tutti fieri del lavoro fatto fino ad oggi. Abbiamo un obiettivo, che nel 2026 il ministro Fitto assicura sarà raggiunto. L'Italia *post* PNRR sarà un Paese più competitivo, non solo per effetto degli investimenti del Piano, ma anche per le riforme e le nuove procedure di spesa che esso ha introdotto. L'Italia in Europa ha sempre più voce; la nostra autorevolezza non è più in discussione grazie ai rapporti internazionali e alla saggia direzione del presidente Meloni. Il Governo ha dovuto fare i conti con un contesto internazionale problematico e sfidante che sta gestendo influentemente. Grazie al nostro contributo nel settore dell'agricoltura comunitaria, come nel caso della PAC, grazie al nostro lavoro sulla valorizzazione del *made in Italy*, uno dei fiori all'occhiello che in Europa porta in dote il Governo Meloni è proprio la *governance* del PNRR. Il ministro Fitto, da solo un anno e mezzo a guida del Dicastero, ha portato il nostro Paese, nell'ambito degli Stati membri, ad essere quello che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I progetti procedono con un'accelerazione oggettiva: basta guardare i dati del 2023, quando sono stati spesi 21 miliardi rispetto ai 24 miliardi complessivi dei due anni precedenti. L'Italia è il primo Stato membro dell'Unione europea a chiedere la quinta rata del PNRR. Insomma, il dato è talmente positivo che smaschera sul nascere qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica. Fatevene una ragione: stiamo facendo bene, l'Italia sta crescendo, siamo competitivi in Europa, siamo tornati grandi nel mondo, determinanti in politica estera ed anche i fondi del PNRR ad oggi sono stati spesi bene e la previsione è spenderli tutti al meglio. Ministro Fitto, il Paese la ringrazia, quest'Aula la ringrazia per la gestione e l'intera *governance* del Piano. Lo stesso Governo, ne sono certa, le è grato per il contributo indispensabile che questo decreto

Presidente del Consiglio, 1.800 euro di *cachet* come compenso per un intellettuale che presta il suo ingegno per parlare del 25 aprile sono troppi.

si può fare. *(Applausi)*. Gli amici giustamente vanno ricompensati per i loro servigi e Brunetta è stato davvero un valente servitore, perché, dopo aver smontato il salario minimo per i comuni cittadini, ha garantito per sé stesso il salario massimo. un capolavoro e siete riusciti a infilare questa porcheria nel provvedimento in discussione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. La vostra parola d'ordine, però - e qui ve ne va reso merito - è erodere. Avete cioè imparato che gli attacchi frontali vanno evitati quasi ad ogni costo, tranne quando sbracate e diventa inevitabile; non parlate più di secessione e di federalismo, perché la gente si mette paura, allora parliamo di autonomia differenziata, così nessuno capisce di che cosa si tratta, che cos'è, ma otteniamo ugualmente la secessione dei ricchi. È fantastico.

modificato, però il Presidente della Repubblica diventa sostanzialmente il maggiordomo del Presidente del Consiglio eletto, come non si vede in nessun'altra parte del globo terracqueo. *(Applausi)*. Agite in maniera obliqua, non diretta, così le persone non si mettono paura.

c'entra niente, voi date autorizzazione ai vostri Presidenti di Regioni di spalancare le porte dei consultori alle associazioni

sponsorizzate in maniera martellante una legge, che è diventata legge di iniziativa popolare ma che viene anche inserita come mozione in molti Comuni amministrati dalla destra, che ha un nome molto romantico, «un cuore che batte», presa pari pari dall'Ungheria del vostro amico Orbàn e riportata in Italia. È una legge di tortura che vorrebbe obbligare le donne che vogliono abortire ad ascoltare il battito del feto.

mandando in televisione a parlare personaggi surreali che ricoprono anche ruoli importanti, che si permettono di definire l'aborto, ossia una legge dello Stato italiano, un delitto e un omicidio, dando quindi a tutte le donne che hanno fatto ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza delle assassine. Questa non è una legittima opinione, questo è gravissimo. *(Applausi)*. Non so se voi non vi rendiate conto delle parole o facciate finta di non rendervene conto, gravissima e inaccettabile la deriva che avete messo in moto in questo Paese. Il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, ieri ha partecipato alla protesta delle associazioni contro questa deriva, per riaffermare il diritto alla libertà e all'autodeterminazione di tutte le donne italiane e oggi parteciperà alla stessa protesta indetta dai sindacati, perché voi oggi avete i numeri, ma non potete vincere nel Paese, perché il Paese non è con voi su questo.

e penso davvero che questo Paese abbia bisogno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma gli obiettivi e i tempi sono stati così stravolti che non voteremo questo decreto su cui state ponendo la fiducia. Noi pensiamo e abbiamo pensato a un piano che ci desse l'opportunità, uscendo dalla terribile crisi vissuta con il Covid, di affrontare alcuni nodi strutturali del nostro sviluppo, in particolare quegli obiettivi trasversali che riguardano i giovani, le donne e il Sud. È un'eredità grande che avete ricevuto dagli altri Governi che state stravolgendo e nello stesso tempo è l'unica leva che avete di crescita, come dimostra questo DEF vuoto che ci avete consegnato. In questo decreto c'è un taglio complessivo delle risorse pubbliche, che si spostano verso il privato, e c'è un taglio rispetto al Sud, penso ai 5 miliardi presi dal Fondo di coesione e sviluppo, che non c'è garanzia che torneranno, non c'è nessuna trasparenza su quel 40 per cento di risorse che dovrebbero andare al Mezzogiorno. Ci sono vincoli su cui il Governo non risponde. C'è una mancata trasparenza sul PNRR.

ospedaliera, fondi che le Regioni avevano impegnato e che non si capisce come ritorneranno su quei progetti. C'è, appunto, un taglio della spesa sanitaria. Su altre tematiche vediamo deleghe in bianco; e poi

un emendamento che non c'entra nulla con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come hanno sostenuto anche l'Unione europea e la portavoce agli affari economici dell'Unione europea. La tentazione è ogni volta troppo forte, lo hanno detto altre mie colleghe intervenendo in quest'Aula: siccome non si può attaccare una legge che funziona, una legge che ha garantito il ricorso all'aborto sicuro, che soprattutto è sopravvissuta a *referendum* e a boicottaggi continui, si cerca di aggirarla, di svuotarla, di boicottarla, appunto, e soprattutto si cerca di stigmatizzare e di colpevolizzare le donne che vi fanno ricorso. Lo fate dove governate, dove già ci sono queste associazioni che pagate anche, come in Piemonte (tra l'altro, per una sorta di eterogenesi dei fini, questo emendamento non vi consentirà di pagarle come fate in Piemonte), lo fate dove non consentite che l'aborto farmacologico con RU486 sia fatto in *day hospital*, come le linee guida nazionali sostengono. Qual è il punto? Parliamo, Parliamo, se ce lo consentite, di che cosa significa l'interruzione volontaria di gravidanza e di qual è la questione centrale. Perché c'è un sapere delle donne, un'esperienza delle donne che oltretutto ha imposto questa grande discussione nel dibattito pubblico, perché fino a cinquant'anni fa era nella clandestinità e nella morte per clandestinità *(Applausi).* Quindi se c'è qualcuno che rivendica la rilevanza politica ed etica di aver posto la questione sono le donne e il femminismo. C'è un sapere di cui non si tiene mai conto, prova ne sia «Porta a porta» e tutti gli uomini a discutere di aborto. Parliamone, perché il tema vero che la 194 riconosce è la centralità della scelta femminile in materia di maternità, sessualità sessualità e aborto. Non è un caso che quella stessa legge parli di tutela della maternità e non si può usare quella parte contro l'altra. Bisogna affidarsi all'autonoma coscienza delle donne. Questo è il punto. Il PNRR lo faceva lo faceva in altro senso: introduceva vincoli come quelli per l'occupazione femminile, introduceva degli obiettivi, come quelli per i servizi educativi 0-6, che andavano nella direzione dell'*empowerment* femminile perché è lì che bisogna andare se si vuole prendere sul serio la questione della maternità e della denatalità, perché siamo un Paese in cui c'è uno scarto enorme tra figli desiderati e figli effettivamente realizzati, perché mancano i servizi, ma anche il rispetto per le donne, perché i figli

sono derogati, non solo quelli sui servizi, ma la gran parte degli appalti: il 62,79 per cento dei bandi sono fatti in deroga a quella norma sull'occupazione in un Paese dove il 55 per cento delle donne non lavora. Chiederete: cosa c'entra questo con la 194? C'entra moltissimo, perché il tema è la piena cittadinanza delle donne e la piena responsabilità e integrità delle donne nel prendere decisioni sul proprio corpo. Non a caso il Parlamento europeo, seguendo l'esempio francese, ha votato una risoluzione che parla dell'integrità della persona e, in questo senso, del diritto a un accesso all'aborto legale e sicuro come un diritto di rilievo costituzionale, è un *habeas corpus* femminile e a questo bisogna guardare, al grande rispetto per la scelta femminile e alla fine di quel potere maritale, medico e della legge che il patriarcato ha segnato sul corpo delle donne. Parliamo di aborto, seriamente, non per stigmatizzare e criminalizzare. Per le donne il tema è sempre stato una questione di soggettività: maternità come scelta,

la legge non si riesce ad applicare, perché il 100 per cento dei medici sono obiettori. Bisogna riconoscere la competenza femminile nel mettere al mondo le persone, gli esseri umani. La prima e l'ultima parola spettano a loro. Su questo le donne sono mobilitate. Quell'emendamento mette in discussione questo: la decisione delle donne. Noi siamo con quelle donne che sono state in piazza ieri e che saranno in piazza oggi al Pantheon. Non vi consentiremo di metterle sotto accusa, non vi consentiremo processi, non vi consentiremo e non vi consentiamo di chiamarle

quest'Aula che c'è poco spazio per il dibattito e che bisognerebbe avere più tempo per parlare e poi si vedono i banchi, soprattutto quelli dell'opposizione, drammaticamente vuoti, come se il dibattito

di tante cose, tranne che del PNRR. Abbiamo sentito parlare di autonomia differenziata, di premierato, di monologhi RAI, addirittura di personaggi surreali nelle trasmissioni TV; abbiamo sentito parlare del DEF, come anticipo forse del dibattito di domani. di domani. Si è parlato poco però di PNRR. Forse se ne è parlato poco perché, al di là delle chiacchiere, poi contano i numeri. Ebbene, i numeri sono 121.000 progetti in corso di realizzazione,

e che il Parlamento, a suo tempo, ha avuto meno di un giorno per poter parlare, esaminare e approfondire le centinaia di pagine di articoli, grafici e formule che il PNRR prevedeva. Oggi si fa polemica su questo? Si fa polemica perché qualcuno rivede obiettivi irraggiungibili (scritti in maniera irresponsabile, magari per poter dire, come sempre, che l'Italia fondi europei), per metterli a sistema, per far sì che questi miliardi che arriveranno vengano spesi nell'interesse della collettività, e se alcuni obiettivi vengono rivisti, vengono rivisti non perché si tagliano i fondi, ma per far sì che quei programmi e quei progetti vengano effettivamente realizzati, spostando su altri punti del nostro bilancio e della nostra legislazione le misure che serviranno. C'è una polemica che è stata fatta sull'emendamento che riguarda la legge n. 194 e io la voglio affrontare con totale chiarezza, perché poi si parla sempre e si legge poco. Io voglio leggere l'articolo 2 della legge n. 194, non l'articolo 1.123, il secondo articolo della legge. Tale «I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base

L'emendamento afferma che le Regioni organizzano i servizi consultoriali, nell'ambito del PNRR, e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. alla maternità. Qual è la differenza tra questo emendamento e il testo reale della legge? Qual è l'attacco alla legge n. 194? Qual è l'attacco al diritto delle donne ad abortire? Dove sta, se non nel fare ovviamente assoluta polemica basata sempre sul nulla, perché non si sa come attaccare il Piano nazionale di ripresa e di resilienza che il Governo sta portando avanti? Questo è il tema. Bisogna stare attenti, quindi, a non generare nel Paese momenti di odio ingiustificato,

Questo è il motivo per cui è stato presentato tale emendamento, che non mette in discussione nessun diritto, nessuna legge e non crea nessuna modifica. Di questo stiamo parlando. Attenzione allora a seminare odio nel Paese, soprattutto quando questo è assolutamente ingiustificato. Parliamo di questo; e se proprio dobbiamo tirare fuori temi che non c'entrano nulla con il PNRR, parliamo di quello che, insieme al PNRR, il Governo sta facendo e dell'immagine che l'Italia sta avendo in Europa e nel mondo. Lo sta dicendo non certo un giornale conservatore inglese come "The Telegraph", che dice che l'Italia della Meloni sta facendo ciò che la Gran Bretagna poteva solo sognare di fare; l'Italia sta diventando invidiabile e nel PIL supera Gran Bretagna, Spagna, Francia e Germania. Lo aveva già detto "The Economist" a gennaio, ribadendo questo concetto. Vogliamo parlare dei soldi recuperati a mo' di record dell'evasione fiscale? 31 miliardi, mai successo prima. Vogliamo parlare del record occupazionale e della bassa disoccupazione che c'è nel nostro Paese? Anche questi sono dati mai registrati prima. Vogliamo parlare della riduzione del *deficit*? Parliamo di questo, non di polemiche che avvelenano il Paese, che mettono in discussione diritti che non sono mai stati messi in discussione e che danno una linea chiara e di indirizzo preciso di questo Governo alla nostra Nazione. Qualcuno dice anche che il Paese

perde, se vogliamo, come Presidente in Sardegna, ma voi sapete che le liste di centrodestra in Sardegna hanno superato abbondantemente i risultati delle elezioni politiche. Io non so se il Paese non è con noi; sicuramente non è con nessun altro e forse, però, il lavoro che stiamo facendo è davvero apprezzato.

in cui il Governo giustamente presenta un decreto-legge con cui vuole portare all'approvazione le ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e invece

se da un lato lo comprendo, dall'altro dico che però è colpa sua ed è colpa di questa maggioranza. Cosa c'entrava la riforma della legge n. 194 con questo emendamento sul PNRR? Cosa c'entrava? Io ancora non l'ho capito e nessuno me lo potrà spiegare, perché davvero è ultronea, come si suol dire in diritto, è una materia che non c'entrava nulla.

per dire basta a provvedimenti di urgenza e basta a provvedimenti nei quali vengono inserite norme eterogenee ed ultronee, che non c'entrano niente, se non è bastato questo a evitare che venisse inserita, nel dibattito parlamentare alla Camera, una norma di modifica della legge n. 194 dentro le disposizioni che vogliono garantire un'efficace attuazione del PNRR, se non è bastata la parola autorevole del Presidente della Repubblica, chi mai potrà riuscire a farvelo capire? Chi ci potrà riuscire? *(Applausi)*.Penso proprio nessuno, perché, se non basta il Presidente della Repubblica, francamente nessuno di noi qui ha l'ambizione o la convinzione di essere più autorevole di lui. Quindi, con tutto il rispetto, evidentemente ci dobbiamo in qualche modo rassegnare a stare attenti a queste manovre che succedono nel passaggio tra la Camera e il Senato, in cui i testi che presentate, nominati, come in questo caso, urgenti per l'attuazione del PNRR", sortiscono poi altre disposizioni che non c'entrano assolutamente nulla. E non mi si venga a dire che era necessario introdurre nel PNRR la norma che prevede la facoltà per le Regioni di avvalersi delle organizzazioni del terzo settore per sostenere la maternità. Non me lo si venga a dire, Ministro, perché con il PNRR sono stati tagliati i fondi per la sanità. *(Applausi)*. Vogliamo sostenere le donne? Vogliamo sostenere la maternità? Ci mettevamo i soldi, ci mettevamo le risorse e facevamo un percorso; davamo gli strumenti per garantire alle donne che sono in difficoltà, alle ragazze madri, ma anche alle donne di fascia d'età più alta, di avere un sostegno. Avevamo a cuore questo? Facevamo un altro percorso, non certo l'ingresso ad associazioni del terzo settore non meglio identificate, che devono dare un sostegno alla maternità. Ma già nei consultori il sostegno alla maternità viene dato, già l'assistente sociale nel consultorio c'è, già lo psicologo c'è, già la legge prevede il colloquio con lo psicologo per la donna che vuole sottoporsi all'interruzione volontaria di gravidanza. Non è che dovevano arrivare le associazioni del terzo settore *(Applausi)* per farci sentire il battito del feto e farci distogliere dall'insano intento. Diciamocelo francamente, l'obiettivo è questo, ed è ciò che già si fa nella Regione Piemonte. Forse una piccola modifica effettivamente la vedo, perché nella Regione Piemonte le organizzazioni *pro-life* hanno ricevuto un pagamento per la tortura

erogato soltanto se hanno almeno due figli, perché uno solo non basta; non parliamo poi se si tratta ad esempio di donne che non riescono a portare a termine una gravidanza: in quel caso non c'è nessun sostegno, né psicologico né economico. *(Applausi)*. Vogliamo dire che questa è una norma a sostegno della maternità? Vogliamo ancora andare avanti con questa retorica? Penso che sia meglio accantonare l'argomento; però non possiamo accantonare la questione, perché è davvero grave. Questo testo di legge viene portato all'esame del Senato impedendo ai senatori di svolgere qualsiasi attività. In 5a Commissione bilancio non sono stati non sono stati neanche discussi gli emendamenti, perché sono arrivati questa mattina e non c'era il tempo. Infatti il provvedimento arriva in Aula senza il mandato al relatore. Lo spiego per chi ci segue: significa che questo testo transita dalla Camera così come è stato approvato e arriva al Senato blindato; nessuno di noi ha la possibilità di apportare alcuna modifica, né noi dell'opposizione né i senatori della maggioranza. Peccato però che la Costituzione preveda altro: prevede un sistema bicamerale in cui entrambe le Camere legiferano, entrambe le Camere fanno emendamenti, entrambe le Camere votano gli emendamenti e modificano il testo.

Camera mentre al Senato bisogna accettarli *obtorto collo*, in silenzio, zitti, senza poter dire nulla e senza poter fare neanche un dibattito. Questo infatti non è un dibattito, ma diventa o rischia di diventare una discussione oziosa, nella misura in cui qualsiasi cosa noi diremo non servirà a modificare il testo di legge, non servirà neanche a indurre una riflessione nella maggioranza, se lo vogliono modificare, perché non potrebbero ritirare l'emendamento neppur

testo apodittico: significa che il Governo ci rappresenta una situazione economica e noi dobbiamo dire che ci sta bene così, perché tanto non abbiamo neanche una tabella di riscontro dei numeri. Siamo all'apoteosi del dibattito parlamentare impedito totalmente. Signor Presidente, mi rendo conto che il testo meriterebbe un articolato confronto, un dibattito, un esame approfondito, perché il PNRR è decisamente ed inequivocabilmente l'unica risorsa presente in bilancio, l'unica risorsa sulla quale si programma la spesa, poiché non ce ne sono altre. E allora, riceviamo un testo dal quale dipende anche la nostra proiezione economica di crescita, quello che pensiamo o immaginiamo di poter raggiungere in termini di PIL. Lo portiamo in Aula, impediamo il dibattito dobbiamo limitarci a recepire questa normativa urgente, così dichiarata, così definita, con la quale, in sostanza, il Governo vuole razionalizzare la spesa e distribuire meglio le risorse. Avevamo già visto, nel corso del precedente anno, che le risorse che erano state destinate ai Comuni per i piani di rigenerazione urbana erano state tolte dal PNRR, ma sempre in maniera fumosa. Noi non abbiamo una stretta corrispondenza fra risorse, spese e progetti irrealizzati. Nella relazione questi dati mancano. La stessa Corte dei Conti ha rilevato questa fumosità nella relazione del Ministro. Distribuire le risorse e poi fare un monitoraggio della spesa: queste potevano essere le tre linee guida di questo testo di legge. Razionalizzare, distribuire, monitorare: poteva anche andare bene, almeno in senso generale, dire che queste risorse, queste disposizioni, servivano a raggiungere questi tre obiettivi. Questo, però, se il Governo, come sempre, non rinuncia al suo approccio centralista e statalista. È inutile continuare a dire che si punta sulla autonomia differenziata, che si vogliono responsabilizzare le stazioni appaltanti, che si vuole dare una maggiore speditezza alla spesa. maggiore speditezza alla spesa. Non è così perché, come sempre, il Governo coglie l'occasione per creare nuove figure centraliste. Abbiamo l'unità di missione dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assorbe il personale e le risorse dell'Agenzia di coesione. Poi abbiamo le cabine di coordinamento che sono deputate alle prefetture, uffici territoriali governativi che devono occuparsi di monitorare le stazioni appaltanti, nella misura in cui queste sono sostanzialmente gli enti locali, per verificare che sappiano spendere. Poi abbiamo questa figura, ormai mitologica per questo Governo, che sono i commissari. I commissari sono la soluzione a ogni problema, secondo il Governo. Ne abbiamo uno che si occuperà di Ne abbiamo uno che si occuperà di verificare che siano portate a casa le misure per realizzare gli alloggi universitari; uno che si occuperà del recupero, dell'utilizzo e della valorizzazione dei beni confiscati alla mafia e uno con un compito, ancora più incredibile e creativo, per il contrasto agli insediamenti abusivi nello sfruttamento dell'agricoltura. Questa è davvero l'apoteosi della visione centralistica di un Governo che non si fida delle autonomie locali, che ha deciso di depotenziare la spesa, di togliere risorse alle stazioni appaltanti quando sono enti locali e progetti che erano già stati finanziati, che toglie le risorse alla sanità, che crea cabine di regia come se fossero cabine degli stabilimenti balneari ed è convinto che così il PNRR verrà portato a casa. Complimenti.

Questo è il dato fondamentale.

siamo impossibilitati a fare una discussione, a presentare un emendamento, a introdurre una modifica o ad abrogare qualche parte. Siamo praticamente chiamati a dire un sì o un no. Questo è il fatto fondamentale. C'è lo svilimento del ruolo dei parlamentari, di questa Aula parlamentare, e questo è inaccettabile, anche perché noi ci troviamo di fronte a un Piano che è clamorosamente in ritardo. Nello stesso tempo si è definito un *omnibus*, dove si è messo più o meno di tutto. Ora, questo piano doveva sì affrontare il problema delle disuguaglianze. Questo è il dato fondamentale. Noi abbiamo avuto una serie di risorse maggiori rispetto ad altri Paesi,

strutture. L'ultima relazione del Governo indica 42,9 miliardi di uscite del PNRR cumulate a fine 2023, valore decisamente inferiore rispetto a quello che era previsto addirittura nella NADEF del 2022.

dal punto di vista della struttura produttiva, guardando soprattutto alla transizione ecologica, dando quindi un impulso fondamentale in questa direzione, mi chiedo dove siano questi piani e dove sia questo dato. Questo è il problema. Questa è la critica che mi sento di fare e di sottolineare. troviamo invece - parlo anch'io di questo problema - un emendamento sul pro-vita. Ora, francamente, dovreste avere il coraggio, visto che siete un Governo politico, di affrontare i temi per quelli che sono.

che ha una rilevanza morale e politica fondamentale: affrontiamola per quella che è; abbiate il coraggio di discuterne nel Paese e alla fine,

possa cercare di contribuire? In tutto questo impedite ai senatori e alle senatrici di contribuire in tale direzione. Pure alla Camera avete dovuto almeno recepire una norma importante, importante, perché sul PNRR, sulla questione del lavoro e della sicurezza, avete speso quasi niente fino a oggi: questo è un dato e purtroppo questa è la situazione.

è inutile girarci intorno - il fatto che molto spesso succedono incidenti mortali, in particolare plurimi, per i problemi della catena degli appalti e dei subappalti, quindi in sostanza del ciclo produttivo, che

perché bisogna fare una discussione e anche affrontarla, perché dopo che si è discusso bisogna agire: non è facile dire alle imprese (che magari sono microimprese distribuite sul territorio) come fare rete e come costruire un modello organizzativo in grado di

Questo è il dato fondamentale. Rispetto a tutto ciò c'è bisogno di un confronto, di una discussione e poi di una sintesi. La maggioranza ovviamente prende anche decisioni e nessuno gliele può negare,

patente a punti. Io avrei molte cose da dire: non sono contrario, sono d'accordo, ma avrei molte cose da dire, perché se si fa la patente a punti, per cui l'unica previsione è sostanzialmente quella di

vi appassiona poco. Signora Presidente, oggi avrei voluto illustrare un ordine del giorno, ma poiché siamo ad oltre 50 fiducie, chiaramente non ci sono più né emendamenti né ordini del giorno: tutto è decaduto, perché ormai in questo Parlamento non si discute e non ci si confronta. Il Parlamento è diventato esclusivamente il luogo di propaganda di questo Governo e temo che purtroppo continuerà ad esserlo fino fino alle elezioni europee. È un luogo in cui costantemente vengono utilizzate armi di distrazione di massa: anziché parlare di quanti pochi fondi abbiamo speso di quelli stanziati per il PNRR; anziché dire che il Paese è fermo; anziché dire che la produzione industriale è in calo da undici mesi; anziché dire che ci sono 5,7 milioni di poveri che aspettano di essere aiutati dalla politica; anziché dire che ci sono quattro milioni di italiani che ormai hanno rinunciato a curarsi, questo Governo oggi ha deciso di tendere la mano agli antiabortisti e farli entrare nei consultori, perché questo è diventato l'argomento della discussione. Presidente, avrei voluto presentare un ordine del giorno di cui ero molto fiera, perché era il frutto del lavoro compiuto all'interno dell'intergruppo che mi onoro di presiedere, presiedere, che si occupa di diritti fondamentali della persona, un luogo di democrazia partecipata in cui oltre 100 cittadini si riuniscono anche qui in Senato, una volta al mese, per costruire proposte a tutela dei diritti di tutti. seduta plenaria che facemmo a gennaio, ci occupammo del tema della violenza di genere, all'interno del quale rientra anche la violenza riproduttiva,

Presidente, ci siamo occupati di questo tema nell'intergruppo perché c'è un *report* della Commissaria europea per i diritti umani che a dicembre 2023 ha espresso grande preoccupazione per gli ostacoli che oggi in Italia incontrano le donne che vogliono sottoporsi ad interruzione volontaria di gravidanza. Questi ostacoli sono riassunti in dodici punti, ma ne elenco solo alcuni. Le liste d'attesa sono lunghissime: le donne, in alcune Regioni, devono aspettare anche un mese per potersi sottoporre all'interruzione volontaria di gravidanza; manca l'attuazione delle linee guida del 2020 sull'aborto farmacologico nei consultori: sono moltissime le Regioni che ancora non le seguono e addirittura addirittura da nove Province le donne devono trasferirsi per sottoporsi all'interruzione volontaria di gravidanza e in Basilicata una donna su tre deve andare fuori Regione.

*(Applausi)*. Con quell'ordine del giorno, quindi, volevamo chiedere proprio di implementare tutti i percorsi per permettere a tutte le donne su tutto il territorio nazionale di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ma volevamo anche chiedere un monitoraggio costante e qualitativo dei dati che oggi non c'è, con un osservatorio permanente. Oggi quel monitoraggio lo fanno le associazioni, i centri d'ascolto e quella rete che si è creata nella società civile per sostituire ciò che lo Stato avrebbe dovuto fare in questi cinquant'anni, da quando è stata approvata quella legge, e ancora non ha fatto. Anziché rispondere a queste criticità rilevate dalla Commissione europea, che cosa fa questa maggioranza? Apre le porte dei consultori alle associazioni antiabortiste e addirittura prova a giustificare quest'apertura dicendo che tutto sommato era già prevista nella legge n. 194. Vi chiedo, allora, se era già prevista, perché avete dovuto fare un emendamento. Poi prova anche a giustificare tale scelta dicendo che queste associazioni aiuteranno le donne a superare gli ostacoli socioeconomici: per superare gli ostacoli socioeconomici non basta di certo un pacco di pannolini regalato da un'associazione antiabortista. *(Applausi)*. Servono politiche di *welfare* adeguate, l'aumento dei salari e gli asili nido, che invece state tagliando nel PNRR; serve rafforzare la sanità pubblica, che state definanziando; serve aumentare l'occupazione femminile, che soprattutto al Sud è ancora bassissima; serve forse anche il congedo di paternità, di cui invece non volete parlare. Certamente questa norma che avete inserito con un emendamento non aiuta a superare lo stigma sociale che ancora accompagna chi sceglie nel nostro Paese di abortire, nonostante - vi do una notizia l'aborto sia stato depenalizzato come reato nel 1978: vi prego quindi di informare anche la vice direttrice del TG1 che l'aborto non è un delitto, ma è stato depenalizzato. Le chiedo solo un minuto, Presidente, e concludo. La vostra è una proposta anacronistica, perché parallelamente ci sono Paesi come la Spagna o come la Germania che addirittura hanno approvato leggi per tenere le associazioni antiabortiste lontane dai consultori, mentre noi andiamo nella direzione opposta. Peraltro, è una materia totalmente estranea a questo decreto, tanto che ve l'ha dovuto ricordare anche la portavoce della Commissione europea che il provvedimento si occupa di *governance* del PNRR e le associazioni antiabortiste non c'entrano niente. Chiudo ricordandovi un paio di cose. In primo luogo, i consultori sono luoghi laici della sanità pubblica. Vi ricordo anche che quest'Aula è un luogo laico di uno Stato democratico e - fatemelo dire, visto che siamo alle porte del 25 aprile e non tutti riescono a pronunciare questa parola - di uno Stato laico e antifascista. In questo luogo laico che è il Parlamento, noi abbiamo il dovere di scrivere leggi che tutelano tutti i cittadini. Poi, sono i cittadini a scegliere se avvalersi o no di quel diritto. Non provate a mettere in discussione le motivazioni soggettive per le quali una donna decide di portare avanti

da medico, ma non sono rilevanti, né per noi, né per voi, perché quella donna sta solo disponendo del proprio corpo e della propria vita e, nel farlo, non è vincolata a rispondere alle aspettative di nessuno, tantomeno alle vostre. *(Applausi)*.

di modernizzarsi e di intraprendere una strategia per essere competitivo con gli altri Paesi europei. Questo dev'essere il *focus* della giornata: dobbiamo cercare di concentrarci su un'opportunità.

è di metterli in relazione tra di loro, affinché possano concorrere alla crescita del Paese. Oggi anche in 5a Commissione abbiamo discusso soprattutto del perché del perché non possiamo apportare modifiche al provvedimento e del perché c'è stata una sola lettura alla Camera. Ecco, c'è una risposta molto semplice dal mio punto di vista e si chiama tempo, quello che, quando è stato sottoscritto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato ridotto. Ricordiamo infatti che le risorse devono essere utilizzate entro giugno 2026 e quindi

le semplificazioni che sono state previste per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi la semplificazione per quanto riguarda tutte le norme riferite alle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Italia ha una peculiarità derivante da territori bellissimi e diversi tra loro ed ha la specificità di una competenza industriale, artigiana e turistica che necessita di interoperare per poter esprimere la propria eccellenza. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza offre l'opportunità di raggiungere quest'obiettivo. La dinamicità del Governo e del Parlamento deve però poter essere unita nel concorrere a portare a questo risultato, intervenendo anche e soprattutto per raggiungere l'obiettivo. Ricordo che le risorse sono in parte a fondo perduto, ma in grande misura in prestiti che saremo chiamati a rifondere con gli interessi. Gli interventi devono essere quindi mirati e ben ponderati. Ci siamo sempre impegnati a garantire la copertura di tutti i progetti e oggi con questo provvedimento diamo concretezza a tali impegni, trovando la copertura per intero a tutti i progetti che in una prima fase erano fuoriusciti dal PNRR. PNRR. Ricordiamo che, anche quando sono state inserite queste opere, tante di esse sono state tirate fuori dal cassetto, magari nella strategia di mettere in interoperabilità tutte

La rimodulazione del Piano ha permesso di destinare le risorse, perché bisognava anche rimodularle e cercare di metterne anche sul REPower EU. Ricordo che nel REPower EU, quando è stato fatto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, non erano previste risorse in questo capitolo.

un credito di imposta del 45 per cento rispetto alle spese che sosterranno per efficientare gli impianti. Noi diciamo alle aziende italiane che vogliamo investire sull'efficientamento delle loro attività di impresa che, se aumentano la loro efficienza del 10 per cento, gli investimenti che avranno utilizzato per raggiungere quel grado di efficienza saranno loro rimborsati fino al 45 per cento. Ed ecco che, anche qui, la legge di bilancio che prevedeva sostegno alle famiglie per mantenere il loro potere d'acquisto e il Piano nazionale si conciliano, cercando di di dare risorse importanti alle aziende affinché il nostro Paese possa rimanere sempre competitivo.

sicuri. Non esiste: prima della rimodulazione, le risorse erano all'incirca 15 miliardi di euro; alla fine della rimodulazione, le risorse continuano ad essere 15 miliardi di euro; cambia casomai la fonte di finanziamento e da questo punto di vista andiamo su norme già esistenti relative all'edilizia sanitaria. Questa non è un'operazione di taglio, con la quale invece accertiamo e garantiamo al Paese e alle altre istituzioni locali di portare a termine quegli interventi. Tantissime parole sono state spese, anche dal senatore Magni, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro: è stata appunto inserita la patente a punti nei cantieri edili. Nei lavori in Commissione alla Camera gli emendamenti della Lega hanno specificato cose importanti, cioè che tutte le imprese dovranno avere la patente a punti, ad eccezione di quelle che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. intellettuale. Sempre grazie ad alcuni emendamenti del nostro Gruppo, si è introdotto il principio che alle imprese che rispettano determinati criteri, definiti da un decreto ministeriale, potranno essere riconosciuti ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale. Il decreto-legge nel suo complesso interviene anche nella lotta al lavoro nero, con norme più chiare e sanzioni più importanti;

viceversa aiutarle e lo facciamo con una decontribuzione totale per le tante famiglie che decidono di assumere un assistente familiare per occuparsi dei loro anziani: anche questo è un tema che non possiamo sottovalutare, essendo appunto l'Italia uno dei Paesi che stanno invecchiando di più. Va anche ricordata la relativa semplificazione dei regimi amministrativi per le imprese artigiane, prevista da questo decreto-legge. Semplifichiamo infatti i regimi amministrativi di 45 tipologie di attività artigiane: artigiani edili, carpentieri, muratori, allestitori di *stand*, *graphic designer*, imbianchini, ma anche sarti, vetrinisti, ceramisti, creatori di articoli di bigiotteria e così avanti. Gli oneri amministrativi a carico di queste attività verranno ridotti in modo decisivo, arrivando a eliminare il titolo abilitativo per l'avvio delle attività (risparmi burocratici che si tradurranno in risparmi medi di oltre 2.000 euro). Quando pensiamo al nostro Paese, spesso pensiamo in grande, ma poi ci ritroviamo nella vita reale ad aver

meno. In questo provvedimento cerchiamo di dare risposte un po' a tutte le categorie, intrecciando - come dicevo prima - la legge di bilancio con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché vi dev'essere una strategia, quella di un Paese che deve crescere, deve correre e deve diventare competitivo,

doveva permettere all'Italia di recuperare terreno e speranze, dopo il drammatico tracollo economico determinato dal Covid. Doveva servire a riqualificare l'assistenza sanitaria, a strutturare la transizione ecologica, energetica e digitale, a rafforzare la pubblica amministrazione, a preservare e valorizzare l'ambiente come casa comune, anche nell'interesse delle future generazioni, com'è scritto in Costituzione, ad aiutare la generazione dei più giovani europei (italiani, meridionali), nonché a costruire un futuro migliore per tutti, dopo i drammi arrivati dalla pandemia. Invece carenze, ritardi e criticità di vario grado sono elementi distintivi del Governo Meloni nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Da quando il Governo di centrodestra si è insediato, abbiamo assistito a troppi scivolamenti di scadenze. Inoltre, abbiamo visto forti divari, non solo territoriali, nella partecipazione ai bandi di questo piano, con gli enti locali più piccoli in grosse difficoltà e le Regioni del Sud in forte affanno. Abbiamo poi registrato una rimodulazione delle risorse del PNRR priva di criteri obiettivi e di correttivi che potevano servire ad aiutare i territori più disagiati e bisognosi di interventi. Abbiamo annotato, nel contesto, l'ulteriore centralizzazione operata da lei, ministro Fitto, che si è distinto per l'allungamento dei tempi e la confusione prodotta. Riporto qualche dato in maniera significativa. Posto che i progetti ammessi al Piano sono circa 220.000 e che poco più di 1.000 non risultano selezionati e finanziati, stando all'ultimo aggiornamento di fine 2023 risultavano erogati quasi 45 miliardi di euro. Questo significa che nei prossimi tre anni vanno spesi oltre 151 miliardi; in sostanza, oltre il triplo di quanto fatto finora. Secondo il monitoraggio di Openpolis, il Ministero delle infrastrutture guidato dal ministro Salvini risulta il soggetto più indietro, poiché ha ancora 34 miliardi di euro da spendere e ha la quota più alta di fondi attribuiti. attribuiti. Oggi, in fase di conversione, ci ritroviamo pertanto a dibattere di un provvedimento nato tardi e male, Ministro, che non pone alcun rimedio agli errori già fatti dal Governo, dal Governo, che continua a tenere gli occhi chiusi, senza accorgersi della direzione del Paese, dei gravissimi problemi di spesa di questo Piano e delle conseguenze nefaste delle sue scelte. Le domande che ci poniamo, signor Ministro, sono le seguenti: lei è proprio convinto che il PNRR stia andando bene? È consapevole che il suo Governo, fallendo sulla spesa di questo Piano, gioca sulla pelle dei cittadini e su quella delle future generazioni? Ha idea, Ministro, di cosa comporteranno i ritardi in corso per l'economia generale, per il diritto alla salute, per il processo di transizione verde, per la velocizzazione delle pubbliche amministrazioni e per il futuro del Paese, soprattutto per i più giovani? Siamo in tanti, signor Ministro, a credere che lei sia sempre più chiuso nelle sue idee, al punto da non riuscire a cogliere più l'entità dei problemi, la gravità dei ritardi e l'inadeguatezza assoluta di questo decreto-legge sul PNRR. Tra l'altro, se non bastasse, riguardo a questo provvedimento la Corte dei conti si è espressa in termini negativi, decisi e pesanti, che il Governo ha respinto e si rifiuta di cogliere. Secondo la Corte dei conti, il previsto taglio di 1,2 miliardi per gli interventi sanitari colpisce l'equità nella distribuzione delle risorse tra le diverse Regioni. Tale taglio poi penalizza particolarmente il Sud, mette in pericolo l'accesso alle cure dei cittadini e incide pesantemente sulla qualità dei servizi erogati. In pratica, si vanno a colpire gli investimenti regionali già avviati, con l'effetto di rinviare l'attuazione dei progetti a quando ci saranno le risorse disponibili. È un fatto di una gravità inaudita, di fronte al quale purtroppo va registrato il silenzio dei Presidenti di alcune Regioni del Mezzogiorno, che hanno la sanità in ginocchio, gli ospedali fatiscenti, un'assistenza territoriale a terra e un'emigrazione sanitaria alle stelle; stanno però zitti solo per una questione di colore politico. Tutto questo è inaccettabile. Potrei fare l'esempio della Calabria e anche di altre Regioni. La Corte dei conti ha altresì avvertito che il nuovo modello organizzativo previsto in questo provvedimento potrebbe determinare una confusione gigantesca nelle amministrazioni locali, che già non sono state aiutate ad affrontare i problemi legati al PNRR. Tra l'altro, sul piano organizzativo vi sono forti dubbi sul commissariamento previsto per la realizzazione delle opere, atteso che appare totalmente disancorato disancorato da un percorso di meritocrazia e di comprovata specializzazione dei commissari che vanno scelti. Non sono presenti nel dettaglio informazioni sui costi. Infatti, nello specifico, secondo la Corte dei conti, sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie previste andava fatta un apposito elenco. In sostanza, la Corte dei conti ha rilevato la necessità di fugare i dubbi circa la futura necessità di integrazione degli stanziamenti di spesa. È un ulteriore vizio di questo Governo: fare le cose senza una chiarezza sui conti, come se non fosse indispensabile, soprattutto in questo caso, in cui si tratta di gestire e finanziare risorse straordinarie, quanto enormi. Insomma, la situazione del PNRR è preoccupante. Se dovessi sintetizzare non solo quanto ha detto prima, ma anche quali sono i quali sono i punti di caduta più drammatici rispetto a quello che state facendo o no, li sintetizzerei in due grandi criticità. La prima è il grave ritardo e la seconda è la mancanza totale di trasparenza. Il ritardo è dovuto al cambio della *governance* che avete imposto e alla revisione del Piano che avete fatto e che non ha risposto in termini di qualità e di efficienza ad accorciare i tempi, ma semmai li ha aumentati. al secondo elemento di criticità, questo Parlamento non è in grado di conoscere la situazione del PNRR in tempo reale. Questa è una mancanza di trasparenza drammatica. È preoccupante, signor noi siamo molto preoccupati. Anche il vostro silenzio su questo ci preoccupa e impensierisce anche gli amministratori. che diversi osservatori, università ed enti pubblici, hanno interamente mollato il PNRR e non ne controllano più lo stato di avanzamento? Sa per quale motivo? Per la mancanza di dati aggiornati. I tecnici, gli enti privati e le università hanno totalmente abbandonato il PNRR. Ormai per loro è una strada morta, perché non riescono a studiare i dati in tempo reale. Nessuno li conosce. Tutto questo per noi è inaccettabile e tutti questi argomenti, chiari, innegabili e pesanti, mostrano che il Governo ha fallito clamorosamente nell'attuazione del Piano, tradendo le aspettative degli italiani, alimentando confusione e ritardi, ma soprattutto acuendo i divari territoriali. Per questo motivo, siamo fortemente contrari alla conversione di questo decreto-legge, certi invece che un atteggiamento diverso e la condivisione dei problemi con il Parlamento, con gli enti locali, con le autonomie locali e con i tanti amministratori probabilmente avrebbero portato avrebbero portato a risposte positive e a buoni risultati. Invece, probabilmente il tema vero è che al Governo interessa soltanto il potere per il potere, ma, in questo caso, il vostro atteggiamento e comportamento sono politicamente imperdonabili.

ricordando gli investimenti aggiuntivi, pari a circa 25 miliardi di euro, che poi vengono definiti. Ora, negli interventi che mi hanno preceduto, non ho sentito tanti colleghi parlare di questi 25

Invece, tanti altri Comuni, che magari non hanno neanche operato le assunzioni necessarie affinché si potesse andare avanti con le progettazioni del PNRR, non hanno neanche presentato progetti realizzabili, in quanto il Governo di allora, che mandò in Europa tutti i progetti di Comuni e

sento solo tante critiche, ogni volta che si presenta nelle nostre Commissioni e nella nostra Aula, che a me sembrano costruite ad arte e che tante volte sono senza alcun tipo tipo di fondamento. Questo è il mio secondo intervento sul PNRR. Anche in occasione del primo, però, sentii solo critiche: una cantilena e una litania di critiche e considerazioni che nulla che nulla hanno a che fare con la realtà dei fatti e di quello che questo Governo sta facendo su una progettualità voluta da altri Governi. L'importante in questo momento, per una certa parte politica, è demonizzare, in una continua campagna elettorale

che questo Governo abbia messo mano a un provvedimento fatto da loro e che lo abbia in qualche modo migliorato. Ricordo che un collega del MoVimento 5 Stelle, in un'altra seduta d'Aula, utilizzò l'argomento dei banchi a rotelle

potranno raccontare all'Italia la grandiosità di questo Piano, che non è finita nel momento in cui sono arrivati i soldi, ma continua con l'azione di questo Governo. Il "quanto" lo voglio ancora ricordare, caro Ministro e caro Presidente, perché ancora oggi ci dimentichiamo che sono 62,9

ringrazio chi ci ha preceduto come Governo che è riuscito e ha scelto di prendere tutti questi soldi. È stato il Governo giallorosso, il Conte 2, "Giuseppi", chiamiamolo come vogliamo, ma non è stata bravura, perché esistono dei criteri oggettivi e inequivocabili - se qualcuno studiasse, li troverebbe in maniera molto semplice - che spiegano come mai l'Italia ha potuto scegliere di prendere tutti questi soldi nella maggior parte - ripeto - a debito, a prestito. Quindi, come dicevo prima, solo quando riuscirete a metabolizzare il quando, il come e il perché riuscirete a raccontare la grandiosità di ciò che ci può essere quanto bene possono fare al sistema Italia tutte le progettualità effettivamente realizzabili sul nostro territorio italiano, grandiosità che vogliamo salvaguardare. Ed è per questo che il ministro Fitto in maniera incessante e periodica ha cercato di avere un dialogo sempre costruttivo con il Parlamento. Il Governo dovrebbe lavorare sui progetti PNRR e con le norme non si risolvono i problemi: l'ho sentito dire a un collega proprio oggi in Commissione. Grazie, lo sappiamo che con le norme non si risolvono i problemi e ci fa piacere che, come per i banchi a rotelle, abbiate compreso che finalmente i problemi non si risolvono con le norme; non lo è stato per la povertà - lo sapete bene - e non lo sarà per la natalità. Quindi, quando qualcuno ci accusa che in questo accusa che in questo decreto-legge noi, in maniera sarcastica, abbiamo cercato di risolvere il problema della denatalità, ci accusa male, perché lo sappiamo da subito e da sempre che con le norme non si risolvono i problemi che sono ormai atavici. Povertà e natalità sono due problemi atavici che l'Italia ha e che dovrebbero vederci collaborare per la loro risoluzione. I decreti servono per raddrizzare un qualcosa che oggettivamente è stato scritto di fretta e lo sapete anche voi, perché probabilmente in tanti di voi, come quelli che di noi erano all'opposizione allora, quel decreto che istituisce il PNRR non l'avete letto; è stato scritto anche male, come sapete anche voi, e non sarebbe andato avanti. Correggere il PNRR ci ha portato ad essere i primi in Europa a incassare le rate e a operare le rendicontazioni dovute; nessuno della minoranza in questi mesi ha mai avuto un sussulto di dignità nel dire che un pochino ci eravamo riusciti. Non avete fatto mai una parola. Vi do un suggerimento, per il suo tramite, Presidente: controlliamo tutti noi, perché credo che molti cittadini, sicuramente i portatori di interesse, lo facciano in maniera

caro Presidente, sempre per il suo tramite: che tutti gli interventi previsti dai fondi PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. Tanti progetti che sono stati presentati allora, quando non c'eravamo noi,

dei consigli, di fare bene, di fare meglio assieme a voi e oggi lo facciamo in maniera convinta. Quelle risorse sono importanti per il sistema Italia. Una finanziaria, quando viene presa, va spesa bene ed è quello che stiamo facendo grazie a Fratelli d'Italia e al Governo Meloni. io ho terminato il mio intervento sul PNRR. Le chiedo solo un secondo di tempo, perché da donna mi sento di dire una cosa. Sappiamo anche noi che una donna che sceglie di abortire soffre tanto; sappiamo anche noi che si fa quella scelta con il cuore pesante e che il proprio cuore viene lacerato e non permetto a nessuno, a nessuna donna e nessun uomo, di insinuare il contrario. Ho però il cuore e la mente per pensare che ci possa essere sempre un'alternativa, perché non l'ho vissuto sulla mia pelle, ma l'ho vissuto sulla pelle di tante mie care amiche. Per questo sarò al fianco, nello stesso modo, con la stessa faccia, con la stessa forza, con lo stesso amore, ad una donna che ha deciso di fare quella scelta e a una donna che quella scelta decide di non farla. È per questo motivo che voterò convintamente il provvedimento

Signor Presidente, ringrazio innanzitutto i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, sia della maggioranza che dell'opposizione.

questioni che sono state sollevate anche rispetto all'utilizzo o meno delle risorse, alle scelte che il Governo ha fatto rispetto all'utilizzo delle stesse. Lo farò a partire da una considerazione: capisco la

ai quali ho ascoltato le stesse critiche alla Camera. Dico questo perché ciò non vuol dire non aver avuto la possibilità di intervenire nel merito del decreto-legge, di poterlo modificare, di potersi confrontare per più ragioni: in primo luogo perché il dibattito e il confronto c'è stato in uno dei due rami del Parlamento, in secondo luogo al contrario di quanto detto in alcuni interventi, il confronto c'è stato in più direzioni, a partire - lo dico al senatore Irto, che poc'anzi esprimeva delle critiche su questo fronte

proprio rispetto ad una delle questioni fondamentali, che è l'articolo 1 del presente decreto-legge, ha espresso un parere favorevole. Lo dico perché penso che sia importante, come approccio sul PNRR e anche come approccio sul decreto-legge in esame e sui futuri provvedimenti, che ci sia una valutazione più attenta. infatti mettere insieme alcune grandi questioni che sono state oggetto di grandi polemiche, di grandi critiche, con dichiarazioni roboanti nei confronti del Governo e con dichiarazioni molto dure che hanno animato il dibattito politico del nostro Paese per mesi. Per esempio, si diceva che era una follia irresponsabile e impossibile revisionare il piano quando Giorgia Meloni, che non era ancora Presidente del Consiglio, lanciò questa esigenza sia per i problemi di carattere esterno (penso alle vicende collegate all'invasione dell'Ucraina), quindi al grande tema dell'aumento del costo dell'energia, così come all'aumento del costo delle materie prime, che oggettivamente incidevano stravolgendo i contenuti e gli obiettivi del Piano. Mi riferisco anche, ad esempio, al fatto che all'interno della revisione del Piano abbiamo

dicendo due cose che non corrispondevano alla verità. La prima era una polemica strumentale, che sollevava polvere inutile rispetto al fatto che noi avevamo garantito, nonostante l'entità delle risorse da recuperare, che mai avremmo trovato, che avremmo certamente coperto le risorse dei Comuni che erano stati finanziati nel PNRR, e lo abbiamo fatto. L'articolo 1 ve lo dice in modo molto chiaro; e l'ANCI esprime una soddisfazione perché in questo lavoro il Governo ha garantito per intero la copertura degli interventi che per molti mesi sono

C'è stato chi, se non sbaglio la senatrice Bilotti nel suo intervento iniziale, ancora una volta ha - come capita spesso - enfatizzato il grande merito dell'avvio del Piano. Io penso che sia importante ancora una volta, e lo farò ogni volta che verrà sollevato questo pseudo-merito, ricordare quello che è alla base del Piano, ovvero che i criteri in base ai quali il nostro Paese ha ottenuto queste risorse non sono merito di nessuno, sono i criteri dettati dal Regolamento che una lettura di quelle che erano situazioni economiche del nostro Paese e quindi l'aumento o meno del prodotto interno lordo (l'Italia, dopo il Covid, aveva i peggiori dati), l'aumento o meno del tasso di crescita occupazionale (anche sotto quell'aspetto l'Italia aveva i peggiori dati) e il numero degli abitanti. In più, il nostro Piano è così grande per un'altra ragione - lo diceva poc'anzi la senatrice Zedda ed è molto importante sottolinearlo - che è relativa alla dimensione del Piano: 68 miliardi a fondo perduto e 122 a debito, perché l'Italia, insieme alla Grecia e alla Romania, a differenza di tutti gli altri Paesi europei, ha chiesto e preso al 100 per cento le risorse a debito, compiendo un'operazione che è quella che ha visto il Piano assumere queste dimensioni, alle quali sono stati aggiunti altri 30 miliardi di euro di Piano nazionale complementare, che sono stati, anche quelli, presi a debito. Noi quindi, a fronte di oltre 220 miliardi di euro di Piano Piano nazionale di ripresa e resilienza con il Piano nazionale complementare, ne abbiamo oltre 150 a debito e di questo penso che vada tenuto conto in tutte le considerazioni che facciamo sia rispetto all'attuazione del Piano, sia rispetto a ciò era contenuto all'interno del Piano. Lo voglio ricordare perché all'interno dei 122 miliardi di euro a debito 68 erano riferibili a progetti in essere, cioè a progetti finanziati precedentemente al Piano e quindi spostati dentro al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno costituito di fatto uno spostamento di debito pubblico, che erano stati finanziati già con leggi di bilancio precedenti e che quindi non sono stati finanziamenti aggiuntivi, ma che avevano una caratteristica, ovvero quella di avere al proprio interno una serie di elementi, ad esempio il

da una scelta che non era corretta, cioè quella di aver inserito una serie di progetti che non potevano essere nel PNRR, sia perché non sarebbero stati mai rendicontati con le regole del PNRR, sia perché quelle risorse non sarebbero mai state spese nei tempi e nei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Possiamo discutere quanto vogliamo, ma questo è un fatto così così gigantesco ed evidente che non è discutibile rispetto alle opinioni e alle polemiche politiche. Lo dico perché non solo lo conferma l'ANCI, alla luce dell'operazione completata con questo decreto, con il suo parere favorevole, ma anche qui vorrei inserire un elemento. Ascolto molte critiche che sono rivolte al Governo, al sottoscritto, alla maggioranza, e va tutto bene, ma non è che noi abbiamo iniziato un percorso autonomamente e che non abbiamo

con un elenco di inesattezze, sulle quali adesso puntualmente darò delle risposte, che vengono utilizzate a fini più esclusivamente politici che nel merito delle questioni. Noi su questo giochiamo anche un dato reputazionale del nostro Paese. La riuscita o meno del PNRR appare talvolta un combattimento, quasi si esulta se c'è un giudizio negativo o un problema, guardando invece a tenere da parte e nascondere gli eventuali risultati positivi. Non è questo un fatto utile. Il rapporto di medio termine dello scorso febbraio della Commissione europea è un altro fatto; magari non piacerà, ma è un rapporto fatto dalla Commissione Commissione europea, dato a dei valutatori esterni, che sancisce con chiarezza che l'Italia ha la *performance* migliore e raggiunto il maggior numero di obiettivi. Di questo non troveremo molto ritorno e risalto sui mezzi di informazione nel nostro Paese, ma è un fatto che ci incoraggia nel lavoro che stiamo facendo. Ci incoraggia altresì il fatto che abbiamo ottenuto la terza e la quarta rata e che stiamo discutendo oggi per il raggiungimento della quinta rata con una verifica degli obiettivi raggiunti e che questo rappresenta un risultato che non è paragonabile a quello degli altri Paesi. Vuol dire che possiamo esaltarci e rallentare? No, vuol dire che siamo sempre in un percorso molto complesso, perché vorrei ricordare che quando ci siamo insediati noi abbiamo fatto un monitoraggio della spesa, visto che si parla sempre di spesa e che si porta il dibattito sulla spesa; il monitoraggio che abbiamo fatto, sulla spesa era su 126 miliardi di euro della precedente programmazione 2014-2020 e dopo nove anni la spesa, dopo nove anni la spesa, i primi mesi dello scorso anno, era del 34 per cento. Quindi, sinceramente, è abbastanza singolare poter ipotizzare, immaginare e verificare che noi abbiamo una situazione nella quale, rispetto all'avanzamento della spesa del PNRR, si possano esprimere queste critiche. Lo dico anche e soprattutto rispetto a dei dati oggettivi, che sono il paragone il paragone della spesa del 2021-2022 con quella del 2023, alla necessità, se vogliamo, di andare a fare una lettura attenta e articolata che andrà fatta anche della spesa del 2021, 2022 e 2023, per evitare che si rivolga una critica alla spesa complessiva, come se essa fosse esclusivamente quella di questo Governo e si omette di fare una valutazione attenta su ciò che accade. Lo voglio dire con una battuta, ma senza voler essere offensivo, anzi assolutamente, alla senatrice Maiorino che ha fatto un attacco all'onorevole Brunetta. Io non ho da difendere l'onorevole Brunetta, ma da ricordare alla senatrice Maiorino che, essendo lei stata senatrice nella scorsa legislatura, ha votato la fiducia del Governo nel quale l'onorevole Brunetta era Ministro e ha votato tutti tutti i provvedimenti che lui stesso proponeva. Era della stessa maggioranza. Quindi, se lei ha qualche doglianza nei confronti dell'onorevole Brunetta, dovrebbe utilizzarla in modo differente, rispetto a questo... Senatrice, le chiedo di lasciar parlare il Ministro, grazie. forte al Governo in riferimento all'onorevole Brunetta. Io mi sono permesso di ricordare alla senatrice che lo ha fatto che lei, che criticava in modo pesante l'onorevole Brunetta attribuendo a me delle responsabilità, aveva votato la fiducia al Governo nel quale c'era l'onorevole Brunetta e i suoi provvedimenti. Solo questo, nessuna polemica o altro.

dalla revisione del Piano. Anche qui voglio tornare su quel punto che ho affrontato all'inizio; la revisione del PNRR ha comportato non solamente la modifica di circa la metà degli obiettivi del Piano, rideterminandoli e rendendoli adeguati, anche qui approvandoli e condividendoli con la Commissione europea e con tutti gli enti attuatori. E, in secondo luogo, abbiamo anche, nell'ambito di quella revisione, previsto delle scelte. ad una delle critiche che il senatore Magni, se non sbaglio, faceva sulla mancanza di attenzione e di strategia rispetto ad alcuni temi, la transizione, per esempio. Ebbene, siccome il nostro Paese, avendo utilizzato inizialmente il debito

del PNRR, ha garantito, con l'articolo 1 di questo decreto-legge, la copertura di quei progetti e ha finanziato, con la rimodulazione di quel Piano, le risorse per la Transizione 5.0, pari a 6,3 6,3 miliardi di euro, cosa che non era prevista. Così come abbiamo previsto, per esempio, altre risorse sull'agricoltura per i contratti di filiera, abbiamo previsto una serie di investimenti in infrastrutture di rafforzamento della rete energetica ed elettrica del nostro Paese, in accordo con Enel, Snam e Terna, abbiamo cioè messo in campo, nella revisione, una serie di scelte che sicuramente sono molto più strutturate e collegate allo scenario nuovo rispetto alla data nella quale era stato messo in campo il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ho ascoltato una serie di critiche sinceramente abbastanza singolari sulla *governance*. La *governance* che abbiamo varato - consentitemi una lettura opposta ad alcune critiche - è una delle ragioni fondamentali che sta consentendo il raggiungimento di questi risultati: esattamente il contrario rispetto alla critica che viene fatta. È una *governance* esattamente speculare a quella della Commissione europea. Non ci siamo inventati nulla di stravolgente; abbiamo visto come funzionava in Europa la gestione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e quindi anche, complessivamente, di questi interventi e abbiamo visto che la *task force* presso la presso la Presidenza della Commissione europea gestiva in raccordo tutte le altre direzioni generali della Commissione europea. Noi abbiamo ricreato esattamente un modello analogo, snello e funzionale, che si interfaccia con la Commissione europea e la cui *governance* ha consentito di riportare in

strutturali del nostro Paese (basta leggere anche qui i rapporti della Commissione europea sulla politica di coesione per prenderne atto) è quello di rendere efficace ed efficiente la spesa delle risorse europee e, soprattutto, di mettere in rete e in linea il punto fondamentale, che è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con le risorse della politica di coesione, in modo che ci possa essere un'integrazione tra i diversi programmi. A tal proposito, vorrei rispondere ad un'altra delle critiche, che è stata fatta se non sbaglio dalla senatrice D'Elia, sul taglio del Fondo di sviluppo e coesione. Anche questo è un tema che io prima o poi aprirei come confronto; forse sarà opportuno immaginare un confronto di merito con il Parlamento. Si contesterebbe, nell'ambito di questo decreto, il fatto che, per una parte delle coperture dei progetti che sono usciti dal PNRR e che hanno trovato altra copertura, noi abbiamo utilizzato una parte di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, pari a 5 miliardi di euro. È vero; ma è vero non solamente perché,

aggiuntivi sul 2021-2027 per l'aumento del costo delle materie prime da assegnare a tutto il Paese; sono 15,6 i miliardi di euro di tagli dell'FSC per cofinanziare e avviare il PNRR. Tutte risorse, pari risorse, pari a 32 miliardi di euro, prelevate dall'FSC sempre con lo stesso criterio e con le stesse preoccupazioni e utilizzate sull'intero territorio nazionale. Io penso che sia opportuno entrare nel merito e fare delle verifiche, anziché fare una critica di carattere genetico. Così come vorrei

È bene ricordare che noi siamo intervenuti sugli asili nido in tre direzioni. La prima direzione è quella di andare a verificare, sulla base delle osservazioni insormontabili che la Commissione europea ha posto, il fatto che la ristrutturazione di asili all'interno dei quali i posti erano già esistenti non potessero essere conteggiati complessivamente sul numero degli asili (cosa che precedentemente era stata fatta). La seconda direzione: siamo intervenuti per verificare nel dettaglio, rispetto alle risorse destinate agli asili e quindi anche ai numeri che sono stati garantiti per 2.600 interventi complessivi nell'ambito degli asili, e per andare a fare un adeguamento del costo delle materie prime. Infatti il costo di un asilo

Terza questione, abbiamo inserito nel decreto-legge Caivano 500 milioni di euro nazionali per poter andare a implementare e finanziare le risorse per gli asili nido, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vorrei anche replicare rispetto al tema dei commissariamenti, che è stato indicato dicendo che noi interveniamo per togliere i poteri a chi deve gestire. Noi abbiamo fatto tre commissariamenti in questo decreto...*(Commenti).*

così magari si ha l'idea complessiva dei 4 miliardi dei quali stiamo parlando. I 500 milioni sono in aggiunta e il Governo ha deciso di metterli sul proprio bilancio per andare a sopperire e correggere gli errori che ha ereditato proprio sul tema degli asili e che sono stati evidenziati dalla Commissione europea.

trovando la copertura, come abbiamo fatto. Vista la *performance* diciamo non eccezionale - per usare un eufemismo - occorreva trovare una modalità di gestione che potesse finalmente avviare e realizzare questi interventi, che vengono da molto prima

misura che ci siamo ritrovati. Non togliamo il potere a nessun Comune, perché è una misura di attuazione del Ministero del lavoro. Individuiamo la figura commissariale perché è l'unico modo per poter operare, vista anche la complessità

di presunti tagli, perché penso che sia importante anche in questa circostanza spiegare il senso del lavoro che il Governo ha fatto. Noi non abbiamo tagliato un solo euro, per la semplice ragione che originariamente il Governo di allora ha preso i progetti finanziati con l'articolo 20 e li ha spostati nel PNRR. Ripeto, ha spostato i progetti dall'articolo 20 all'interno del PNRR. Noi abbiamo semplicemente preso atto della impossibilità di rispettare i tempi del PNRR, tant'è che abbiamo lasciato all'interno del PNRR 900 milioni di euro; nel piano nazionale complementare, dove c'erano 1,240 miliardi di euro abbiamo lasciato 240 milioni. Complessivamente, i 900 milioni del PNRR, più i 240, più gli oltre 2 miliardi che al momento risultano completamente non programmati sull'edilizia ospedaliera - quindi senza alcun intervento di riferimento - coprono e garantiscono l'intero importo. Ci sarà da lavorare con le Regioni e quindi anche il parere delle Regioni sul decreto è positivo, ma condizionato a questo punto: sospeso, ma condizionato su questo punto. Infatti, abbiamo inviato una lettera, a firma del sottoscritto e del ministro Schillaci, ai Presidenti di Regione, per acquisire lo stato dell'arte dei progetti dell'articolo 20, sia finanziati con accordi di programma sottoscritti, sia finanziati con accordi di programma in via di sottoscrizione,

parte non programmata, quelle Regioni che invece hanno programmato e speso al 100 per cento le risorse dell'edilizia ospedaliera. Quindi, troveremo un coordinamento tra le Regioni che devono andare sul PNRR o sul Piano nazionale complementare e quelle che hanno invece ancora una loro disponibilità sull'articolo 20. Complessivamente, le risorse disponibili erano e sono di oltre 3,1 miliardi di euro; quindi, non c'è nessun definanziamento rispetto a quanto previsto all'interno del Piano. Tutti questi aspetti li ho voluto indicare in modo molto chiaro perché, sinceramente, penso che il dibattito sul PNRR dovrebbe essere un dibattito sempre di più nel merito. Noi oggi siamo impegnati, come ricordavo all'inizio del mio intervento, sulla verifica degli obiettivi raggiunti per la quinta rata e sono convinto che questo lavoro molto positivo con la Commissione europea possa concludersi rapidamente. Il raggiungimento e il pagamento della quinta rata rappresenterebbero un altro importante risultato sul percorso del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo al lavoro sugli obiettivi della sesta rata entro giugno di quest'anno e della settima rata entro dicembre di quest'anno. Lo stiamo facendo tenendo in conto anche che il tema che viene spesso sollevato, quello della spesa, è un tema che merita una riflessione molto attenta, su ciò che è accaduto, su ciò che deve accadere e anche su quelle che sono le ragioni collegate alla difficoltà di spesa in alcuni casi. Per questa ragione, con questo decreto noi interveniamo tanto sulla possibilità di accelerazione e semplificazione, quanto su un altro elemento molto importante per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è l'articolo 2 del decreto. Esso tratta un tema molto dibattuto, che è il tema della responsabilizzazione degli enti attuatori. L'idea che alla che alla fine di tutto sia solo il Governo ad essere responsabile, quando la stragrande maggioranza di queste risorse vengono distribuite a tantissimi enti attuatori, non solo Comuni, ma anche aziende di Stato e altri enti attuatori, a mio avviso merita un'attenzione particolare. L'articolo 2 dedica questa attenzione, perché responsabilizza ogni ente attuatore a mantenere fede ai tempi che sono previsti all'interno delle previsioni e degli obiettivi, perché tutti ottengano un finanziamento del PNRR sapendo che quel finanziamento deve rispettare determinate regole, deve raggiungere quei *target* e deve essere realizzato in quei tempi. Quindi, un processo di responsabilizzazione dell'intero sistema istituzionale del nostro Paese non può che far bene a tutti quanti noi, nella prosecuzione di un lavoro che probabilmente troverà anche altre occasioni di verifica e di adeguamento del Piano. Infatti, non sarà questo certamente l'ultimo provvedimento collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché, inevitabilmente, data anche la dimensione del Piano, che abbiamo ricordato prima, è scontato che noi avremo motivi e momenti di intervento costante in questa direzione, per poterlo adeguare e per poter dare delle risposte in questa direzione. Concludo ringraziando tutti coloro i quali sono intervenuti e auspicando che il tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza possa diventare un tema di interesse nazionale, nel senso che sarebbe molto opportuno e positivo che su di esso ci fossero, più che critiche di carattere generico, spesso non corrispondenti al merito delle questioni, dei suggerimenti concreti per lavorare insieme per migliorare

per l'ennesima volta e sono disponibile, come ho sempre detto, non solamente in Aula, ma anche in Commissione, a confrontarci, non sugli *slogan*, ma sul merito delle questioni. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1110, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. nuova finestra"). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Secondo le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. Passiamo

nell'ambito delle misure per l'attuazione del PNRR. Grazie a questo Governo, lo ricordo, è stata messa a punto una revisione del Piano. È stato un percorso di serietà, per il quale va dato merito al ministro Fitto della bontà del lavoro che ha svolto fino ad oggi e svolgerà nel prossimo futuro, che ci ha portato a tagliare traguardi molto rilevanti. La terza e la quarta rata sono state già concesse e finanziate. L'Italia - ce lo dice l'Europa - è il Paese che registra la migliore *performance* sul PNRR, con una spesa pari a 45 miliardi. Siamo l'unico Paese ad aver richiesto, infatti, anche la quinta rata. Abbiamo riformato la politica del Fondo di sviluppo e coesione e il Governo sta proseguendo con questo lavoro che mira ad un raccordo efficace tra i vari fondi. È un lavoro indispensabile, perché - forse qualcuno se ne dimentica - i 122 miliardi di risorse europee sono a debito. In parole povere, sono risorse che vanno restituite e quindi la qualità - ribadisco, la qualità - della spesa non è un dettaglio, ma è un fattore determinante che incide sulla crescita e, di riflesso, può consentire al sistema Paese di rientrare dal debito. Com'è noto, il provvedimento in esame introduce importanti novità, anche in altri settori, che certamente impattano sulla vita dei cittadini, come la riforma della *governance* sulle guide turistiche, la semplificazione per il rilascio dei passaporti, così come quella sulla sanità e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Parliamo poi del digitale, uno dei punti più salienti, che riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con un investimento significativo nella modernizzazione dei servizi digitali pubblici. L'obiettivo verso cui si sta lavorando e si deve continuare a lavorare è sburocratizzare e migliorare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Come centrodestra, da sempre siamo convinti che lo Stato debba essere amico dei cittadini e delle imprese. Il senso di questo provvedimento è proprio questo: credere in una pubblica amministrazione, che guarda ai risultati e non si perde nei mille rivoli della burocrazia. Il digitale, d'altronde, a nostro avviso, può e deve essere l'anello della catena che unisce o avvicina istituzioni a cittadini e imprese. L'altra grande direttrice su cui poggia il PNRR è la transizione *green*. Sono previsti investimenti nel campo dell'efficienza energetica, negli edifici pubblici e privati, ma anche per sviluppare le energie rinnovabili e per promuovere la mobilità sostenibile. Sono misure che contribuiranno non solo a ridurre le emissioni di gas serra, ma anche a creare posti di lavoro. Vengono garantiti - e qui veniamo ai numeri incontrovertibili 12 miliardi per le imprese: di questi 12 miliardi, 6,3 miliardi sono destinati alla Transizione 5.0 del nostro sistema produttivo. La Transizione 5.0 libera risorse per le nostre aziende. Parliamo infatti di una misura che destina fino al 45 per cento del credito d'imposta per gli investimenti negli impianti aziendali che riducano i consumi di energetici di almeno il 10 Altro capitolo che mi sta molto a cuore è l'agricoltura. Al settore primario andranno infatti 8 miliardi (prima erano 5) e ne sono stati aggiunti altri 3. Questa è la prova inconfutabile di quanto l'agricoltura e gli agricoltori siano centrali nell'agenda politica di questo Governo e di questa maggioranza. Gli agricoltori sono i migliori garanti della sostenibilità ambientale. Ieri, infatti, abbiamo celebrato la Giornata mondiale della terra. Sono loro gli angeli custodi della nostra terra. Ricordate quando dall'opposizione dicevano che il Piano non poteva essere riscritto? La revisione del PNRR sembrava fosse qualcosa di irraggiungibile. Invece, grazie all'impegno del Governo e suo, signor Ministro, queste risorse non solo le abbiamo raggiunte, ma sono addirittura aumentate. Ci tengo ad evidenziare questo passaggio: grazie alla revisione del PNRR, l'Italia (non la destra, il centro o la sinistra, ma l'Italia) ottiene il più grande stanziamento economico mai registrato per l'*asset* primario della nostra Nazione. Questa è la differenza tra il movimento dei no e la politica del fare, che si allea con chi questo verbo lo conosce meglio di chiunque altro, cioè l'impresa. Siamo pratici, come gli imprenditori che al mattino alzano la saracinesca per lavorare e dare lavoro, e ci stiamo ostinatamente impegnando affinché si superi lo schema secondo cui per le imprese lo Stato è percepito troppe volte come un nemico, se non da combattere quantomeno da temere. Noi siamo per uno schema sicuramente differente: le imprese devono potersi fidare dello Stato, perché lo Stato senza le imprese (agricole, commerciali, artigianali e industriali) non può - lo sottolineo - creare i presupposti per far crescere il Paese e dare futuro. Tutte le nostre richieste sono frutto di un costante processo di ascolto delle esigenze del mondo produttivo. Il provvedimento in discussione è frutto del lavoro di ascolto e quindi della concertazione con tutti gli attori che, a diverso titolo, ruotano attorno all'ecosistema del PNRR. Il dialogo è stato lo schema vincente anche con gli enti locali, soprattutto quando parliamo di un altro importantissimo capitolo del PNRR, quello sulle infrastrutture. Per questo oggi il modello di *governance* del PNRR può essere l'occasione per mettere a sistema un nuovo modello di efficienza ed efficacia che sia realmente in grado di mettere a terra i progetti nei vari territori. Io credo - e sfido chiunque di voi a dire il contrario - che se un sindaco di sinistra, di destra o di centro ottiene dei fondi per il suo Comune, per la sua comunità, poco importa se al Governo ci sia una compagine di un tipo o di un altro. Questo è il senso più bello di una politica che costruisce e non demolisce; questo è il senso più bello e autentico di una politica che lavora per la comunità e non per agitare una bandiera. Questo Esecutivo ha rimodulato il piano e lo ha fatto conseguendo conseguendo risultati che sono sotto gli occhi di tutti: dalla rinegoziazione abbiamo ottenuto un aumento della dotazione finanziaria pari a 194,4 miliardi, cui si sommano 2,9 miliardi dovuti all'aumento dei contributi a fondo perduto. Nel capitolo infrastrutture del PNRR il ruolo dei Comuni è centrale: questo provvedimento, infatti, rafforza la capacità amministrativa degli enti locali. locali. Valuto molto positivamente anche l'emendamento della maggioranza che ha innalzato dal 10 al 30 per cento del valore dell'opera l'anticipo che il soggetto (cioè il Comune) può chiedere per gli interventi legati al PNRR. Non solo, i sindaci potranno vedere queste somme erogate entro trenta giorni. Tutto ciò rappresenta una boccata d'ossigeno per tutti gli enti locali e, di conseguenza, una buona notizia per i territori. Sanità e politiche sociosanitarie rappresentano un ambito che sta molto a cuore al nostro Gruppo. È un tema su cui serve più che mai fare un'operazione verità, a partire dalle polemiche strumentali e propagandistiche che abbiamo visto in questi giorni Consentire alle associazioni del terzo settore di entrare nei consultori e negli ospedali non è contro la legge, anzi è sancito dall'articolo 2 della legge n. 1978. Nessuno pensa di toccare quella legge, come qualcuno ha detto. Aiutare le donne a scegliere la vita non è un reato; anzi, è un reato mercificare il loro corpo, come si pensa di fare con l'utero in affitto. Nel campo sanitario e medico l'Italia, purtroppo, sconta anni di mancata programmazione. Nel nostro Paese si è registrata, infatti, una carenza importante di medici e infermieri: ad oggi mancano all'appello 30.000 medici

finalmente si volta pagina. Faccio riferimento a un emendamento che elimina il tetto di spesa del personale sanitario oggi vigente. Merita sicuramente un breve cenno l'articolo 31 del decreto-legge in esame, che prevede il concorso per l'assunzione di 716 ispettori tecnici dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è questione di destra o di sinistra, è una battaglia che dobbiamo condurre tutti uniti, senza distinzioni né appartenenze. Il PNRR, quindi, è l'esempio migliore che serve a farci capire quanto sia essenziale oggi l'Europa e che lo è ancora più negli attuali contesti geopolitici e internazionali. I nostri cittadini sanno che il futuro di tutti noi passa attraverso un rafforzamento politico dell'Europa e noi oggi in quest'Aula siamo e rappresentiamo l'Italia che crede in una buona Europa. Proprio per questi motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

Non c'è dubbio su questo, ma è chiaro che non è compito dell'opposizione dire dove il Governo riesce, l'opposizione ha il dovere di far presente dove il Governo potrebbe fare di meglio, questo è il nostro ruolo e questo cerchiamo di fare. Con le norme non si risolvono i problemi, diceva la collega Zedda che non c'è e che apprezzo sempre molto per l'impegno e la passione che profonde nello svolgere il ruolo di senatore, ma non è certo l'opposizione che ha portato in Aula negli ultimi tempi una serie di provvedimenti che forse non erano proprio necessari per la vita del Paese, che sappiamo già regolamentato da una quantità enorme di leggi e forse sarebbe il caso di non approvarne delle altre, ma invece questa è proprio la direzione che ha preso questa maggioranza, per esempio con le questioni del Master Chef o della città capitale della mobilità.

del PNRR si è parlato già molto nel dibattito e non credo che ci sia molto da aggiungere, anche perché il Ministro ha risposto in maniera assolutamente esaustiva. Provo invece inquietudine per un altro aspetto, di cui anche si è parlato, ma che

in maniera imbarazzante la Commissione europea è intervenuta a stoppare, dicendo che le misure relative all'aborto non c'entrano nulla col PNRR. È imbarazzante, ma questa maggioranza e questo Governo hanno portato avanti, attraverso quell'emendamento, il disegno di spostamento dell'asse sociale del Paese, che hanno evidentemente in mente. È un disegno che parte da un revisionismo storico volto a recidere le radici della nostra democrazia, che sono radici antifasciste per motivi temporali, perché risalgono all'epoca immediatamente successiva alla Seconda guerra mondiale. Questo revisionismo passa dall'intolleranza verso il pluralismo e la libertà di stampa alle questioni sociali trattate come un problema di ordine pubblico. Sono tutti tutti aspetti che si sono visti negli ultimi tempi in quest'Aula a proposito di vari provvedimenti esaminati. È un disegno che, come sempre accade in questi casi, in ogni Paese e in ogni tempo, annuncia il suo primo compimento sul corpo delle persone, che viene politicizzato, colpevolizzato, intaccato nella propria sfera più intima, esattamente come accade in quei Paesi dove la democrazia è una formula vuota, dove vige l'autocrazia, proprio quello che noi qui non vogliamo, perché crediamo della nostra democrazia. È ancora più imbarazzante la difesa dell'emendamento che ha provato a fare il Governo, perché con questo emendamento è evidente che si vuole rendere più impervia la strada per l'applicazione della che è una legge che in alcune Regioni è praticamente disattesa per i pochi centri, le poche risorse economiche e il gran numero di medici obiettori. Qualche domanda bisognerà porsi sul perché il numero più alto di obiettori sia proprio nelle Regioni governate dalla destra: non è che magari qualche direttore generale di ASL, qualche assessore alla sanità fa pressioni sui medici, mettendo sul piano effetti e implicazioni per le loro carriere? Noi non lo sappiamo, ma sappiamo che in Regioni come le Marche targate Fratelli d'Italia esercitare il diritto all'aborto secondo le regole stabilite dalla legge è diventato impossibile e molte donne sono costrette ad andare fuori Regione. Abortire non è semplice - è già stato detto - per nessuna donna: per quanto l'interessata possa essere adulta, strutturata, senza dubbi sulla propria scelta, è per lei sempre un momento di enorme sofferenza interiore, diversissima da persona a persona, che andrebbe gestito soltanto con grande cura, rispetto e delicatezza e a questo servono i consultori. Portare nei consultori le associazioni antiabortiste è come portare in un centro vaccinale i rappresentanti dei no vax; significa trasformare i consultori in campi di scontro ideologico, luoghi di giudizio sociale, di colpevolizzazione delle donne nel momento di maggiore fragilità. Per questo i consultori devono restare strutture sanitarie, di servizio pubblico di uno Stato laico in cui non si parli altra lingua che non sia quella della medicina e della scienza. Vogliamo ridurre il numero degli aborti? Allora seguiamo quello che gli studi dicono da sempre, si lavori cioè sulla prevenzione e sull'educazione sessuale. Il sistema scolastico italiano invece non prevede tale educazione e la lascia, quando va bene, a qualche ora di lezione dell'insegnante di scienze, esattamente come trenta Ci occupiamo qui di scuola parlando di voto in condotta, seguendo ancora una volta la logica dell'autorità e della punizione e non quella dell'autorevolezza e dell'accompagnamento nella crescita degli studenti o, peggio ancora, si parla di scuola per proibire che qualche istituto dichiari festa il giorno del Ramadan, come se nella società le persone fossero plastilina modellabile attraverso divieti e proibizioni. Ecco, questi aspetti sono inquietanti e questo state cercando di fare con questa norma sulla pelle e contro il corpo e i diritti delle donne. Per questi motivi quello che sarebbe stato un voto di astensione al provvedimento deve diventare e diventa, per quanto riguarda il mio Gruppo, un voto contrario.

Alle 16,22 lei è intervenuto e ha detto una cosa sacrosanta. Ha detto che il PNRR è una cosa talmente seria che dovrebbe essere oggetto di discussione profonda tra di noi, dovremmo cercare di aiutarci.

Certo, stupisce che io voglia fare un grande dibattito con l'opposizione e poi pongo la fiducia. Il problema è che se vogliamo affrontare il tema del PNRR, bisognerebbe spogliarsi di ogni ideologia. L'ideologia di chi a destra ogni volta ci fa la telecronaca; è arrivata la terza, la quarta rata, sta arrivando la quinta rata. È normale che arrivino le rate. Non ho mai sentito nessuno dire che bello, ho pagato il mutuo. È normale che in un accordo arrivino le rate del PNRR. Allo stesso modo bisognerebbe liberarsi dall'ideologia di chi dice che abbiamo ottenuto 200 miliardi. Hanno dato 200 miliardi all'Italia non perché c'è stata una trattativa del Governo, ma perché c'è stato un algoritmo che ha spiegato che, essendo l'Italia in condizioni peggiori degli altri, aveva uno spazio di maggiore intervento. Liberiamoci dalle rispettive ideologie e guardiamo la realtà per come è. Questi soldi non li abbiamo ottenuti. Li stiamo prendendo a prestito dai nostri figli. È chiaro o non è chiaro che siamo in presenza di un'incredibile montagna di denari investiti sul futuro dell'Italia, vent'anni o quindici, ci chiederanno conto le prossime generazioni? È per questo, signor Presidente, signor Ministro, che io avverto l'esigenza di parlare in quest'Aula del PNRR, nonostante non sia l'argomento che va di moda, anzi, per andare sui giornali c'è bisogno di richiamare questioni etiche. Così come per avere la prima pagina dei giornali, c'è bisogno di aprire un dibattito sull'antifascismo, grazie alla solerzia di qualche funzionario RAI che, a mio giudizio, cerca di fare un favore a voi di destra e non si rende conto di aver fatto il più classico degli autogol,

del gruppo dirigente della RAI, che è riuscito a fare questa roba veramente un complimento lo merita a tutti i livelli. Se facessero così con la campagna degli Stati Uniti d'Europa, se avessero questa capacità di dedicarvi grande lungimiranza e intelligenza, faremmo il 20 per cento. *(Applausi)*. Vengo alla sostanza. Smettetela con la retorica dell'abbiamo ottenuto questi soldi; questi sono i soldi dei nostri figli. Ministro Fitto, ci conosciamo da qualche anno: non faccia la parte di quello che chiede considerazioni puntuali e poi si sdegna se qualcuno fa riferimento al CNEL e al presidente Brunetta. Vede, lungi da me l'idea di difendere una collega dei 5 Stelle sulla vicenda del CNEL, che ci ha visto su parti contrapposte nel referendum del 2016; ma questo PNRR serve a rilanciare il Paese o serve a rilanciare il CNEL? *(Applausi)*. L'idea che voi stiate mettendo dei soldi per il CNEL, signor Ministro, è una barzelletta che non fa ridere. Qui non si tratta di giudicare Renato Brunetta, su cui ognuno ha il suo giudizio (il mio peraltro è storico). Il punto centrale è che voi restituite, con i soldi dei vostri figli, uno stipendio al presidente del CNEL, pur non essendo in presenza dei requisiti che consentirebbero astrattamente lo stipendio, perché si tratta di essere non già in pensione. Andate a violare la legge Madia, andate a fare una norma che viola la legge per dare dei soldi a Renato Brunetta, perché altrimenti non vi sta in piedi il giocattolino. State sprecando i soldi degli italiani in marchette! *(Applausi)*. È diventato un marchettificio il PNRR; avete il coraggio di dirlo, sì o no? Non è così? Diceva un grande artista, Munari, tutti sono capaci di complicare, ma pochi sono capaci di semplificare. Caspita, ma fate le assunzioni per il PNRR! Cioè il PNRR serve a rilanciare il Paese nel virtuoso rapporto con le imprese. Ho trovato addirittura lirica l'espressione di De Poli, vivendo una fase di romanticismo assolutamente suggestiva, laddove ha parlato degli agricoltori come degli angeli custodi. Quando il mio amico De Poli ha questa visione così lirica sugli angeli custodi, io sento battere il cuore. Ma scendiamo scendiamo un po' più sulla pratica e lasciamo per un momento la poesia: avete riempito il PNRR di assunzioni! Come li chiami, De Poli, angeli custodi anche quelli? Ma gli angeli custodi che assumete in tutti i provvedimenti per Lollobrigida a cosa servono? A cosa serve che, in ogni provvedimento che questo Governo porta in Aula, ci sia un'assunzione per Lollobrigida? Allora fate un pacchetto e fategliele tutte insieme, anche se poi ancora non ho capito come mai continuiamo ad assumere gente per Lollobrigida: o per controllargli i treni o per inserire il il formaggio nel menù, perché ha bisogno di gente, o per fare delle dichiarazioni veramente suggestive sull'antifascismo. Per quale motivo continuiamo ad assumere al Ministero dell'agricoltura? La verità è che gli italiani devono sapere che voi state sprecando un'occasione; questo è il motivo per cui votiamo contro. E mettete lo spreco dei soldi degli italiani in scelte che sono ridicole: 60 milioni per la base in Albania, dove andare a portare i migranti, sapendo che ci sono 4 milioni e mezzo per un porto, 60 milioni e mezzo per la base in cui identificare i migranti in Albania. I soldi del PNRR vanno per 65 milioni in territorio albanese, perché voi impiegate 600 milioni di euro per andare ad Abbiamo già avuto una discussione con il ministro Fitto, in un piacevole incontro in una scuola di Maglie (il suo Comune), dove io dicevo che secondo me alla fine, al massimo, i migranti che potranno essere accolti in Albania erano 1.500, mentre il ministro Fitto raddoppiava questa cifra in termini di attese, dicendo che secondo secondo lui sarebbero potuti essere 3.000. Che siano 1.500 o 3.000, 600 milioni di euro dei soldi degli italiani, di cui 60 milioni presi dal PNRR, sono una vergogna. Metteteli nei centri di formazione e fate lavorare questi ragazzi, per dare una mano alle aziende del Nord-Est. *(Applausi)*. Non continuate questo elenco di sprechi, che sta facendo paura. Vado a chiudere. Ce ne sono ancora tanti di argomenti, ma non ho voglia di fare l'elenco finale. Io trovo che questo Governo ci stia prendendo in giro, ministro Fitto; glielo dico con la consueta amicizia e la tradizionale stima che comunque le porto. L'emblema di tutto questo potrei farlo con mille esempi. Oggi ho visto che sui giornali scrivete che volete fare gli 80 euro,

contenti. Si legge che la Meloni vuol fare come Renzi e vuol dare 80 euro agli italiani. Ma se si va a vedere la norma, si tratta di 80 euro *una tantum* per la tredicesima alle famiglie con un bassissimo livello di reddito, laddove gli 80 euro di cui si parlava e su cui c'è il marchio registrato sono 80 euro che per dieci anni sono stati

sugli *spot.* Oggi dite che sono arrivati i soldi del PNRR. Bene, avete preso questi soldi, avete rifiutato il dibattito perché ponete la fiducia, e mettete i soldi per risollevare non l'Italia, ma il CNEL, per pagare non le famiglie, ma Brunetta, per continuare a fare degli *slogan* che porteranno l'Italia ad essere indebitata. Il conto tanto lo pagano le prossime generazioni, che a voi non interessano, perché a voi interessano le prossime elezioni. Felice il Paese in cui finalmente torneremo a pensare alle prossime generazioni e non ai vostri sondaggi e alle vostre elezioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

ai cantieri, se ad esempio faccio il rapporto tra la Lombardia, che è la regione più sviluppate d'Italia, quella che ha il PIL più elevato d'Italia, il mercato del lavoro più consistente, il numero di occupati più alto e le retribuzioni più alte,

siamo in ritardo sul terreno dell'innovazione? Forse sono tanti elementi, ma è il confronto che permette di affrontare e dare delle risposte non propagandistiche. Il dato vero è che ci viene impedito di fare una discussione

una politica di accoglienza diffusa, coinvolgente, formativa, che sia in grado di rendere la manodopera una risorsa, perché questo è il dato fondamentale che dobbiamo attuare. Quindi, una politica di integrazione in grado di non creare allarme, che non deporti le persone in Albania perché, se sono tante e di colore nero, fanno paura ed allora è meglio che stiano lontane dall'Italia. Questo è il dato fondamentale ed il problema è come affrontarlo su questo terreno.

le persone che fanno un lavoro ripetitivo sono le più difficili e le più ostili al cambiamento, perché, ovviamente, il cambiamento fa paura. Faccio un esempio banale, perché bisogna parlarci concretamente.

per le condizioni economiche e normative e per le condizioni dei lavoratori. Bene, allora facciamo così: evitiamo di fare i giustizialisti, ma stabiliamo che, anziché fare tante storie in tutti i tribunali, apriamo una sezione composta di magistrati che si occupano di sicurezza sui posti di lavoro. Lo possiamo fare? Io penso di sì, eviteremmo di fare tante discussioni inutili al Paese il messaggio che il controllo c'è. Questa è la cosa che vi chiedo, questo è il dato fondamentale. Per questa ragione sono contrario a questa impostazione del PNRR. Giustamente qualcuno ha detto non ci state dicendo la verità. State facendo una serie di marchette elettorali. È chiaro che non parliate, perché fare queste scelte vorrebbe dire dare una risposta, magari prima delle elezioni. In questo Paese si vota tutti i giorni e credo che questo non si debba fare. Per queste motivazioni, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente contro

oggi ci troviamo ad approvare, non solo nel corso di questa legislatura, il quarto decreto-legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Io ho ascoltato non soltanto la replica del Ministro qualche minuto fa, ma anche alcuni interventi dei colleghi, in particolar modo dei colleghi dell'opposizione, che hanno lamentato tutta una serie di argomenti che ritengo siano anche fuori tema rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che oggi ci troviamo ad affrontare.

Siamo arrivati al quarto decreto d'urgenza perché sono stati fatti numerosi passi in avanti, sono state già impegnate e utilizzate numerose risorse e poi anche perché il Consiglio Ecofin dell'8 dicembre dello scorso anno ha rimodulato il Piano stesso e quindi oggi il Governo italiano è costretto ad intervenire con una serie di progetti non previsti dal Piano nazionale che avevamo qualche mese fa,

per le complicazioni del nostro Paese - perché il Governo, dal punto di vista economico, sta facendo molto bene - ma per la situazione congiunturale economica che ci troviamo intorno, che condiziona le scelte del Governo. Ecco perché oggi è importante snellire la procedura amministrativa prevedere ulteriori strutture, se utili a spendere tutti i soldi, perché il compito che ci siamo imposti in questo Parlamento e come Governo è riuscire a spendere tutti i 200 miliardi di euro che, come dicevo, servono anche allo sviluppo del nostro Paese.

Ho letto anche tutta una serie di interventi delle categorie che oggi vengono toccate da questo decreto e tutte hanno espresso grande soddisfazione, soprattutto la categoria degli enti locali. Voglio dirlo in quest'Aula, da pugliese: l'ANCI stessa si è espressa in favore del decreto-legge al

tenute in seria considerazione anche per i progetti che - come qualcuno diceva in quest'Aula - sono stati definanziati e che verranno ulteriormente compresi. Per questo le categorie che sono state coinvolte e che entrano nel decreto-legge in esame hanno espresso soddisfazione per la sua approvazione.

alla ricerca, alla digitalizzazione, alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, agli investimenti infrastrutturali, ai trasporti e agli enti locali.

Altro elemento positivo è l'aumento del 30 per cento delle anticipazioni per tutti gli interventi, che è proprio diretto a risolvere quei problemi anche economici e di liquidità che hanno molte amministrazioni comunali. Infatti, chi è stato amministratore comunale sa quante difficoltà ci sono nell'utilizzare risorse che

il ministro Fitto non è più in Aula e quindi non può ascoltare qualcosa che avrei preferito potesse ascoltare direttamente, ma andiamo avanti. Non vorrei tornare sulle modifiche apportate alla legge n. 194, perché ne hanno parlato estesamente e molto bene le colleghe del mio Gruppo che mi hanno preceduta, ma lasciatemi dire una cosa, perché da questa maggioranza si vedono inviti al liberismo più sfrenato quando si tratta di temi economici, ma

Certo, è difficile pensare che da quella parte si possa levare un grido di aiuto o in difesa dell'autodeterminazione delle donne, se le colleghe di maggioranza si fanno appellare al maschile e ci tengono molto, a partire dalla presidente

Evidentemente, però, la cultura patriarcale e maschilista probabilmente permea talmente tanto le donne della maggioranza, che forse pensano di doversi mascolinizzare per contare qualcosa e fare strada nei loro partiti. Ma torniamo al decreto-legge in esame. Rimango sempre su uno dei mantra che tanto piacciono alla Presidente del Consiglio: voler lasciar fare a chi vuole fare, per tornare al liberismo di cui sopra. Peccato che, nel caso del PNRR, quelli che vogliono fare liberi da qualsiasi vincolo e controllo siano furbetti e delinquenti che vogliono essere liberi di fare come gli pare, tant'è che recentemente proprio la procura europea ha dovuto denunciare che ci sono stati 600 milioni di euro di maxitruffe sul PNRR proprio in Italia tra il Veneto e altri Paesi, cioè di 206 inchieste a cui stanno lavorando in merito al PNRR ben 179 riguardano l'Italia, l'86 per cento. Che dire? È un *record* di cui andare fieri, non c'è dubbio. E pensare che, secondo voi, non c'era bisogno di fare particolari controlli, tant'è che avete abolito il controllo concomitante della Corte dei conti, vi apprestate con altri provvedimenti ad abolire l'abuso d'ufficio, chiedete solo un intervento e l'azione del Comitato antifrodi, invitandolo ad occuparsi del PNRR (come se ci fosse bisogno di un invito: secondo me, dovrebbe farlo di *default*, ma evidentemente, nell'ottica di questa maggioranza, l'idea di controllare che qualcuno non rubi vale solo quando si tratta di superbonus e reddito di cittadinanza). Torniamo a noi. Fino ad ora è stata messa a terra una percentuale quasi irrisoria nei primi quasi quattro anni di questa misura. Arriviamo addirittura solo all'8 per cento, togliendo quello che è stato speso per Transizione 4.0 e superbonus, misure derivate dai Governi precedenti. Senza di quelle, il tiraggio ad oggi e la messa a terra di queste ingenti risorse per il nostro Paese sarebbe un numero da prefisso telefonico. Che fate, pensando di poter risolvere il problema? Accentrate tutto, quando all'inizio avete preteso e imposto una *governance* che fosse diffusa e non accentrata a Palazzo Chigi, perché il Governo Conte voleva accentrare tutto in mano sua e controllare tutto; chissà che imbrogli volevano fare quelli del MoVimento 5 Stelle, noti alle cronache per truffe, imbrogli, latrocini *(Applausi)*, acquisto di voti, compravendite e cose varie. Infatti, le cronache dei giornali ne sono piene tutti i giorni, neanche fossimo un Fratelli d'Italia qualsiasi. E invece, avete preferito una *governance* diffusa. Appena siete arrivati voi al comando, vi siete resi conto che forse così non funzionava bene e che forse volevate controllare un po' meglio, alla luce, quella sì, della vostra grande esperienza in questi settori, quindi avete pensato bene di accentrare tutto nelle mani del ministro Fitto (che mi dispiace non sia qui), a partire dalla cabina di regia del PNRR, alla ZES unica, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione, e va bene così. tutto in mano a lui, abbiamo fatto una sorta di Ministero dell'economia-*bis:* forse perché Fitto e Giorgetti non vanno tanto d'accordo? C'è qualche dissidio tra il Gruppo Lega e il Gruppo Fratelli d'Italia? Chissà, ce lo domandiamo. Il risultato è che non è migliorato proprio niente, perché siamo ancora allo zero virgola. Avevamo così chiesto in un emendamento presentato a questo provvedimento che ci fosse la possibilità di avere una Commissione parlamentare di vigilanza sull'attuazione del PNRR. Va bene tutto, infatti, però questo Parlamento qualcosa potrà ancora contare in questo Paese o dobbiamo farci esautorare da tutto *(Applausi)*, perché tanto i migliori sono tutti al Governo

Naturalmente, qualsiasi proposta passa sotto la mannaia dell'ennesima fiducia. Pensare che alla fine della scorsa legislatura non facevamo altro che sentire urlare

Però, naturalmente, qualsiasi problema in questo Paese è colpa del superbonus, di quei cattivoni del MoVimento 5 Stelle che hanno fatto questa misura che - udite, udite - ha fatto scendere il rapporto debito-PIL di oltre il 17 per cento - non so se avete capito bene la cifra - oltre ovviamente ad aver fatto salire il PIL del 13 per cento in due anni, ottenendo, oltre al recupero del PIL negativo dovuto alla pandemia del 2020, un bel rimbalzo e un ulteriore avanzo rispetto agli anni precedenti la pandemia. Chissà come mai negli altri Paesi europei, che pure avevano avuto meno problemi di noi, tutti questi effetti non ci sono stati. Oltretutto, c'è stato un incremento di introiti fiscali di circa 140 miliardi. Lo voglio ripetere: 140 miliardi, questi sì, effettivi e certificati negli ultimi anni. Probabilmente non saranno proprio tutti merito del superbonus, ma una buona parte parrebbe proprio di sì, a fronte di soli soli 41 miliardi effettivi di esborso per crediti, che sono stati riscossi per il

Il ministro Fitto prima ha detto che non è vero che ci sono stati 1,2 miliardi di tagli sulla sanità; peccato che lo smentiscano i suoi stessi Presidenti di Regione, l'intera Conferenza Stato-Regioni e che l'abbia smentito pure il presidente Garavaglia in quest'Aula qualche settimana fa,

tutto questo fa emergere solamente una cosa: la vostra palese incapacità di gestire i fondi del PNRR, che sono arrivati in Italia grazie al presidente Giuseppe Conte. *(Applausi)*. E non parlo dell'ammontare dei fondi, quello sì, stabilito con parametri oggettivi e non casuali. È la stessa esistenza del PNRR ad essere merito del presidente Conte, che è riuscito a combattere i falchi dell'*austerity* e a ottenere una norma solidale. Per la prima volta, l'Europa ha mantenuto fede ai propri principi solidaristici, quelli su cui si fonda, ed è stato solo grazie al presidente presidente Conte. Per tale ragione ci opporremo sempre agli scempi dovuti alla vostra incapacità di gestire questo tesoro, anche dei nostri figli, e voteremo convintamente contro il decreto-legge

di questo tesoro lasciato ai nostri figli e spieghiamo un po' come funziona, perché qua vedo, come sempre,

Praticamente l'unica differenza fra emettere un BTP e il PNRR, quantomeno per la parte debito (che è la principale), è che non stanno immediatamente sul conto del Tesoro, ma l'emissione è da parte dell'Unione europea; dal punto di vista contabile è però esattamente identico, quindi stiamo facendo debito, ossia il fardello per le nuove generazioni, l'orribile debito pubblico e così via (a giudicare dalle solite parole di tutti, quando parlano del debito pubblico), quindi questo non tesoro, ma fardello per le nuove generazioni è tutto a carico nostro. Se uno va sulla pagina del MEF, trova esattamente il dettaglio delle cifre ricevute e delle rate da pagare. Faccio notare, per esempio, che fra pochi mesi cominciano le prime rate per ripagare un altro tesoro, il Sure

il primo semestre del 2025) bisogni cominciare a restituire i soldi arrivati dall'Unione europea. Qual è la differenza fra i due indebitamenti?

delle nostre emissioni; di sicuro, non può essere più basso rispetto alla differenza fra lo *spread* che paga l'Unione europea e quello che paghiamo noi. Stiamo quindi parlando di una differenza che non può essere superiore al punto percentuale. Che differenza c'è, se questi soldi li otteniamo con i nostri BTP oppure con questo sistema bizantino? La differenza, dal punto di vista puramente ragionieristico, alla fine è nulla, perché è evidente che, se emetto BTP, al momento del pagamento delle cedole, già subito una parte, vale a dire il 12,5 per cento, viene recuperata in termini di tasse. Viceversa, per la restituzione all'Unione europea non incassiamo assolutamente nulla. Dall'altra parte, è evidente che, se le emissioni sono come le ultime che sta effettuando il Tesoro, vale a dire quelle mirate ai cittadini italiani (come i BTP Valore), l'interesse viene pagato al cittadino italiano, il quale riceve questi interessi e probabilmente li spende. Nel momento stesso in cui inizia a spenderli, ecco che lo Stato italiano cominciare a incassare soldi derivanti dall'IVA e da ogni altro tipo di tassazione che questa spesa produce e che oltretutto normalmente produce sul territorio italiano, quindi è un rimettere in circolo denaro per l'economia. I tassi di interesse che dobbiamo pagare all'Unione europea sono pagati secchi all'esterno, quindi non incassiamo niente. Dal punto di vista della convenienza ragionieristica pertanto, il PNRR - questo regalo, questo tesoro del presidente Conte - non ci conviene. D'altra parte, continuo a insistere su questo: una cosa negoziata da Conte e Gualtieri vi pare mai che possa essere una gran convenienza? Ma li avete controllati? Dal punto di vista ragionieristico, quindi, non c'è purtroppo niente da dire, non è conveniente. Ci siamo trovati dentro questa situazione e bisogna cercare di gestirla al meglio. Adesso vediamo qual è la differenza fra un'emissione di BTP - abbiamo detto che normalmente ci conviene di più - e quello che stiamo facendo. Mi rivolgo a tutti i miei colleghi che sono intervenuti lamentando l'esautorazione del Parlamento: il PNRR è l'esautorazione del Parlamento.

a spostare quanta più parte possibile di questi soldi da cose inutili, com'era previsto inizialmente dai paletti messi dall'Unione europea, a cose che invece

Mi piacerebbe molto avere decreti omogenei, uno che parla di lavori pubblici, uno che parla di sicurezza sul lavoro, uno che parla di cultura e uno che parla di assunzioni nei tanto contestati Ministeri. Certo, mi piacerebbe molto avere lo scrutinio,

da altri, che è contro il Parlamento. Basta ricordarlo. Arriviamo adesso alla parte dei *grant,* ma vi è anche una parte di sussidi,

ha un lievissimo problema: si sta rendendo conto che, anche per loro, dato che sono saliti i tassi, salgono i costi relativi a questo PNRR. Ogni costo aggiuntivo della parte dei sussidi dunque ripartito esattamente con gli stessi criteri con cui normalmente vengono ripartiti i costi di tutta l'Unione europea, quindi la nostra quota parte, quella che normalmente ci vede pagatori netti, è ripartita esattamente nello stesso modo. nel bilancio dell'Unione europea, quello cui noi partecipiamo direttamente, ecco che magicamente dobbiamo metterci i soldi (e quanto più salgono gli interessi, più ne dovremo mettere). Questa era la parte sui *grant*, vale a dire sui sussidi, quindi non ci sono nessun tesoro

di "eliminazione" della possibilità di controllo del Parlamento su cifre così importanti, cui dobbiamo necessariamente far fronte, perché ci siamo trovati il pacchetto pronto. Apprezzo veramente moltissimo il lavoro del ministro Fitto: se non ci fosse un

ottenuti con titoli di Stato, per poi decidere noi sul momento che cosa fare, anche perché, mentre buona parte di questi obiettivi sono obsoleti, viceversa, guarda caso, le risorse che possiamo ottenere sui mercati finanziari sono pronte per la decisione di tutti. però dovrebbe essere chiaro a tutti, ogni volta che parliamo di PNRR, è di non lamentarci se il Parlamento opera sempre di meno. E stiamo attenti a quando, in futuro, l'Unione europea ci proporrà altre forme di debito, perché le sirene hanno già iniziato a suonare.

Signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico voteremo contro il decreto PNRR per il metodo e per il merito. Ci dispiace farlo, perché sul PNRR abbiamo investito tantissimo con le nostre donne e i nostri uomini migliori, che sono stati artefici del fatto che per la prima volta venisse costruito un piano a livello europeo, finanziato con debito comune, per affrontare le conseguenze del Covid e provare a rilanciare la nostra economia. Lo abbiamo fatto con il Governo Conte II e lo abbiamo fatto con Draghi, convintamente. Mi dispiace dover ricordare al collega Claudio Borghi che il tandem Conte-Gualtieri ha portato più di 200 miliardi in Italia, convincendo la Germania *(Applausi)*, cosa che loro non sono riusciti a fare, perché il ministro Giorgetti, rispetto a quello pensato da Gentiloni,

metodo, un po' tutti abbiamo esagerato - dobbiamo ammetterlo - con l'eccesso della decretazione d'urgenza, ma qui si sta passando il limite. Il Comitato per la legislazione ha scritto nel suo parere cose molto vere sull'eterogeneità. Questo è un decreto che parla dell'attuazione degli investimenti del PNRR: di grazia, che cosa c'entrano l'albo dei periti, l'esonero contributivo per il lavoro domestico, gli interventi per la Pedemontana lombarda e le risorse per l'accoglienza agli ucraini? Tutte cose giuste, ma fate un decreto *ad hoc:* qui parliamo di attuazione del PNRR. Dove la straordinaria necessità e urgenza di inserire qui dentro i fondi per costruire i centri d'accoglienza in Albania, quando ancora non si sa se siamo in grado di farlo? Infatti, ci sono una serie di di approfondimenti da fare per capire che è una cosa da matti spendere 800 milioni per costruire un sistema analogo all'estero *(Applausi)*, duplicando, con aliquote di polizia penitenziaria, aliquote di polizia giudiziaria, magistrati, cancellieri e impiegati, moltiplicando i costi per una cosa che non sarà fattibile. Ancora, quali sono i criteri di straordinaria necessità e urgenza per inserire, a decreto fatto, nella discussione parlamentare, temi legati alla disciplina delle guide turistiche o in materia di Camera di commercio? Poi la chicca, l'arcano: il mistero di dover inserire norme in materia di servizi consultoriali; ma che cosa hanno a che fare con la necessità di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli degli interventi del PNRR, se non per fare una marchetta elettorale sulla pelle delle donne, perché questa è? *(Applausi)*. Voglio dirlo allora in maniera molto chiara: da questo punto di vista, la legge n. 194 del 1978 fu un compromesso alto e un confronto fra diverse culture e sensibilità politiche che si confrontarono a lungo. Qui, in un provvedimento che non c'entra niente si inserisce una norma

ha bisogno di sentirsi accolta, compresa, informata e sensibilizzata, non colpevolizzata rispetto a quello che l'aspetta. Questo è il punto fondamentale, che non capite,

le donne e gli uomini nel momento della costruzione di una famiglia. Ci aspettavamo che fossero inserite invece norme per rifinanziare il bando degli asili nido; ancora, non ne vediamo traccia. Ci si dice che sono stati messi i soldi, ma il bando?

continui a dire che così è stato fatto anche in passato. A noi non interessa; a noi preme che questo Governo dia risposte alle Regioni, che si sono viste togliere 5 miliardi che erano destinati ad altri interventi, per provare per provare a coprire i tagli che sono stati fatti, perché i definanziamenti sono tagli rispetto a investimenti attesi dai Comuni, da amministrazioni locali e da comunità che da tempo aspettavano fondi per lottare contro il dissesto idrogeologico, per la rigenerazione urbana, per le periferie

all'articolo 20 della legge sull'edilizia sanitaria. Tutte le Regioni di tutti i colori, di centrodestra e di centrosinistra, hanno scritto al Governo per dire che quei soldi andavano per altri interventi. Io penso a casa mia, Provincia di Varese, al nuovo ospedale che doveva unire gli ospedali di Busto Arsizio e di Gallarate: i varesini aspettano di capire se verranno tagliati i soldi per quest'ospedale o se verranno tagliati quelli per altri ospedali, per interventi di messa in sicurezza di quelle realtà. È giusto mettere i Presidenti di Regione, di qualsiasi colore politico (in questo caso il Presidente è della Lega), davanti al dilemma

che abbiamo chiamato «Ecosistema innovativo della salute», in cui le innovazioni e gli investimenti nella tecnologia erano ancora più importanti, perché abbiamo visto che durante la pandemia non solo non eravamo preparati perché non avevamo adeguati servizi sociosanitari territoriali, ma non avevamo investito in particolare nel tema delle nuove tecnologie. L'*hub* per le pandemie, il polo di Siena, era un investimento fondamentale. Con la scelta di definanziarlo, di tagliarlo e di stralciarlo, si mette a rischio un investimento fondamentale per la prevenzione su un tema delicato come quello delle pandemie. Io spero che questo Governo ci possa ripensare e trovare le risorse necessarie per mandare avanti un tale progetto. mio intervento su quello che, a mio avviso, è il tema dei temi, che abbiamo posto anche questa mattina in una conferenza stampa come Gruppo Partito Democratico. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse il ministro Fitto, per chiedergli

crescerà il prodotto interno lordo (PIL) e hanno legato quel tendenziale agli investimenti nel PNRR (non ci hanno detto nulla del programmato, quindi domani andremo a discutere di cose che non conosciamo e non sappiamo). però, è a rischio lo stesso tendenziale, perché se non siamo in grado di mantenere gli impegni sull'attuazione del PNRR e siamo in clamoroso ritardo, rischiamo di fare i conti sbagliati sulla pelle degli italiani, perché a quel punto, se non ci sono quegli investimenti, altro che i numeri che ci sono sul tendenziale, rischiamo la recessione per la dabbenaggine di questo Governo che non sta attuando gli investimenti fondamentali sul PNRR. *(Applausi)*. Questa dev'essere l'ossessione del Governo, non altre: non la lottizzazione della RAI, né riforme inutili come quella dell'autonomia differenziata e del premierato. Facciano le riforme che sono contenute nel PNRR per far fare un salto in avanti al nostro Paese.

doverosi da parte non solo dell'Assemblea, ma soprattutto di tutti gli italiani, per il grandissimo lavoro fatto dal Governo Meloni e dal ministro Fitto per non perdere le risorse del PNRR, mettere a terra i progetti e i programmi necessari al rilancio di questo Paese e soprattutto dare una necessaria risposta a quella che è stata dapprima dapprima la crisi pandemica che - lo ricordiamo tutti - ha fatto scaturire la nascita del PNRR, una crisi globale in cui - dobbiamo ricordare anche questo e il Ministro lo ha detto molto bene - le risorse che sono arrivate all'Italia sono purtroppo il sintomo di come l'economia italiana

tutte le risorse che poteva a debito, e sono oltre 150 miliardi. Ebbene, in questi mesi, già da prima, in campagna elettorale, e subito appena si è insediato il Governo, non abbiamo fatto altro che sentire la voce di cassandre che di volta in volta, quasi auspicando una sconfitta non del Governo, ma dell'Italia, dicevano che il Governo era in ritardo sulla terza rata, che i soldi non sarebbero arrivati, che avremmo perso risorse importanti per l'economia del Paese e poi per la quarta rata hanno fatto Ora che siamo invece a smentire con i fatti di volta in volta queste cassandre, non abbiamo sentito neanche una voce che avrebbe dovuto essere di gioia e di orgoglio per il lavoro fatto dal Governo. Queste cassandre e questi gufi sono stati smentiti con i fatti, già a partire dal presupposto per cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza non poteva essere modificato, per cui non potevano essere apportati correttivi, che invece sono stati e sono necessari affinché queste opere possano trovare un'applicazione pratica per il futuro della nostra Nazione. Tale considerazione, che sembra basilare, è stata completamente ignorata da una componente politica, che evidentemente spera, in cuor suo, che l'Italia fallisca e che questi obiettivi non vengano raggiunti. Noi invece, con grande pragmatismo e la grande capacità di non solo gli obiettivi, ma soprattutto le problematiche, abbiamo visto un Governo al lavoro fin da subito, perché è innegabile che la crisi economica e il rincaro dei prezzi e dei costi dovuti alle guerre hanno avuto un impatto pesante su quelle che dovevano essere le risorse e le operatività messe a terra. Nonostante questo - lo dice

in questo modo non si vede un risultato che non è solo per la destra o il centrodestra, ma per gli italiani, cercando di togliere un merito importante per questa revisione e per il lavoro fatto

a dispetto di chi continuava a parlare di fallimenti di questo Governo, certifica invece un risultato completamente opposto. Nessun taglio; lo voglio ribadire perché è necessario fare, a onore di chi ci ascolta, un'operazione verità. allora solo su alcune delle misure perché in quest'Aula oggi si è svolto un ampio dibattito, ma si è parlato veramente poco delle misure del PNRR. Abbiamo 12 miliardi a favore delle imprese, 6,3 miliardi per la Transizione 5.0 8 miliardi per l'agricoltura. Erano 5 e noi abbiamo scelto di investirne ulteriori 3. Non lo abbiamo fatto a seguito delle proteste che giustamente gli agricoltori e gli allevatori hanno fatto contro Bruxelles, ma lo avevamo fatto già prima, consapevoli che questo è un comparto essenziale

dalle polemiche sui commissariamenti, che oggi vede alcune inattività. E allora abbiamo giustamente deciso di intervenire anche con risorse importanti per un problema che riguarda i nostri giovani e il nostro futuro.

riprendo le parole che giustamente ha usato nella sua replica il ministro Fitto. In tema di sanità non ci sono tagli; gli ospedali e le strutture che vengono finanziati hanno trovato un diverso capitolo di copertura finanziaria nell'articolo 20. per un'operazione che non vuole depotenziare e togliere fondi della sanità, ma vuole semplicemente portare a termine quei progetti *(Applausi)*, perché altrimenti nel giugno 2026 quelle opere non sarebbero state completate e avremmo perso i finanziamenti del PNRR che hanno una scadenza temporale ben precisa. Tutti noi abbiamo una storia nei nostri territori e sappiamo quanto siano lunghi gli appalti e le procedure. Questa operazione che è a costo pari, anzi aggiunge risorse alla sanità, è stata fatta per salvare quei progetti e non per cestinarli. Sempre in tema di sanità ho sentito parlare di ma allora qualcuno è contrario che si possano assumere gli specializzandi per dare una linfa importante *(Applausi)* di medici e professionisti sanitari all'interno delle nostre strutture che oggi mancano - ricordiamocelo - per l'assenza di una programmazione e per politiche sbagliate a livello europeo, che hanno visto il personale sanitario come un costo che grava sui bilanci? Ci troviamo oggi così senza medici di medicina generale e senza l'opportunità di avere nuove assunzioni per il personale sanitario e i medici ospedalieri. Qualcuno pensa che questo provvedimento sia un *omnibus* da cassare? Ce lo dica entrando nel merito e non facendo solamente solamente polemica politica. *(Applausi)*. Stessa storia per il fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina. Sono tutti temi che vanno a impattare positivamente su un *vulnus* che abbiamo ereditato e sul quale ci stiamo spendendo.

sapendo di mentire, chi dice che il Governo ha messo mano, ha cambiato e con questo provvedimento sta cambiando la legge n. 194. *(Applausi)*. Noi, coerentemente con quanto detto e fatto, stiamo semplicemente dando piena attuazione alla legge n. 194, voluta dal legislatore, una legge di grandissimo equilibrio e di grandissimo rispetto per le diverse sensibilità che compongono il nostro Paese, ma soprattutto con grande rispetto per quelle donne che si apprestano a fare una scelta in un senso che sicuramente è lacerante per ogni donna che la compie o che pensa di farlo e poi cambia idea. In Italia è garantita

e ne ha fatto, anche in questo dibattito, un uso strumentale e una bandiera politica credo che non abbia reso alle donne italiane un servizio giusto e di rispetto. Vedo che il mio tempo sta terminando e non voglio aggiungere molte parole, se non dare proprio la parola alla legge n. 194, leggendo quello che la legge prevede quello che oggi c'è in Italia e che - lo ribadisco - con l'emendamento e con questo atto non viene assolutamente toccato. *(Applausi)*. Coerentemente con quanto dichiarato, si va ad applicare quanto prevede la legge n. 194. A volte mi stupisco che chi la usa come una bandierina non ne conosca il testo o forse decida di ignorarne alcune parti che invece noi reputiamo essenziali, proprio per garantire la libertà della donna; reputiamo essenziale che ci sia libertà di scelta e che tali parti possono essere applicate. La legge n. 194, all'articolo 2, prevede che

concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita».

1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. estratto a sorte il nome della senatrice Versace).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Versace.

nella quale sono stato eletto e nella quale sono nato, Venezia, che ha un legame storico secolare con l'Armenia e con la comunità del popolo armeno, le cui tracce nel nostro territorio risalgono addirittura ai tempi dell'impero bizantino. Abbiamo un'isola a Venezia, che si chiama appunto San Lazzaro degli Armeni, in onore

Il 24 aprile è una data importante, che molti non conoscono, perché ci sono tante, troppe pagine della storia che non sono state mai scritte o, in altri casi, sono state strappate. Ricorre in quella data la Giornata del ricordo del genocidio degli armeni, il grande male che ha colpito questo antico popolo cristiano durante il primo conflitto mondiale. È di fatto, quello del popolo armeno, il primo sterminio di massa del Novecento. La notte tra il 23 e il 24 aprile 1915 a Costantinopoli iniziarono il rastrellamento della *élite* culturale armena, l'uccisione sommaria e la conseguente deportazione in massa della popolazione nelle zone interne turche dell'Anatolia, con le cosiddette marce della morte, durante le quali, lungo il tragitto, migliaia e migliaia di persone. Questo massacro, condotto dai Giovani Turchi al Governo dell'Impero ottomano, durò, di fatto, fino al 1916. Il movente fondamentale che ispirò l'azione del Governo dei Giovani Turchi fu l'ideologia panturchista, il sogno di un immenso territorio nel Mediterraneo e nel bassopiano turanico e la determinazione a riformare lo Stato su una base monoetnica, linguisticamente e culturalmente omogenea. Armeni, greci, assiri ed ebrei: l'Impero ottomano era costituito, di fatto, da un mosaico di etnie e religioni. La popolazione armena, la più numerosa, di religione cristiana, che aveva assorbito gli ideali dello Stato di diritto di stampo occidentale, con le sue richieste di uguaglianza costituiva un ostacolo al progetto di omogeneizzazione del regime. L'obiettivo degli Ottomani era la cancellazione della comunità armena come soggetto storico, culturale e soprattutto politico. Non secondaria fu la rapina dei beni e delle terre degli armeni, che servì da base economica della futura Repubblica kemalista. La pianificazione del genocidio avvenne tra il dicembre del 1914 e il febbraio del 1915. Come dicevo prima, la notte del 24 aprile 1915, l'*élite* armena che viveva a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, venne arrestata, deportata ed eliminata. Poi si procedette al disarmo e al massacro dei militari armeni, costretti ai lavori forzati sulla linea ferroviaria Berlino-Baghdad. Nella primavera fu dato il via alla deportazione sistematica della popolazione armena verso il deserto di *Deir* *ez-**Zor*. Pochi vi giunsero vivi: la maggioranza fu sterminata nel corso di vere e proprie marce della morte. La quasi totalità degli armeni scomparve dalla terra abitata da più di 2.000 anni e i loro beni furono confiscati. Un milione e mezzo di persone perse la vita, i due terzi degli armeni dell'impero ottomano. Molti furono i bambini islamizzati e le donne inviate negli *harem*. Signora Presidente, è evidente che da parte del Governo turco, nell'immediatezza degli avvenimenti dei primi anni Dieci, non ci fu la presa di coscienza dell'enormità della tragedia che aveva causato la propria scelta politica nei confronti della popolazione armena. Sono passati centonove anni da allora e purtroppo sono pochi gli Stati nel mondo che riconoscono il genocidio degli armeni da parte dei dei turchi. Nel 2015, Papa Francesco, nel ricordare il centenario del genocidio, dichiarò: «Nel secolo scorso la nostra famiglia umana è passata attraverso tre enormi tragedie senza precedenti: la prima, che è ampiamente ritenuta il primo genocidio del ventesimo secolo, ha colpito il popolo armeno». La montagna sacra, l'Ararat, oggi all'interno dei confini turchi, può essere ancora contemplata dagli armeni nel territorio della loro piccola Repubblica sorta nel 1992 dalla dissoluzione dell'Impero sovietico e la vista di quelle cime oltreconfine alimenta quotidianamente negli armeni un sentimento di perdita. Sulla Collina delle rondini a Yerevan, che è la capitale dell'Armenia, il memoriale del *Metz Yeghern* (il grande male), l'Olocausto degli armeni, racchiude ed esprime l'impotenza e l'imponenza soprattutto della tragedia. Per concludere, la situazione nel Caucaso è una polveriera anche oggi. Venti di guerra continuano a minacciare quelle terre ed i popoli che le abitano. È gravoso, ma necessario, che la comunità internazionale operi per garantire la pace in quell'area martoriata e ovviamente anche evitare che terribili eventi come quelli del 1915 possano rinnovarsi.